Signor Presidente, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità negli ultimi due decenni il tasso di obesità in Europa è triplicato: ogni anno un milione di decessi e dodici milioni di anni di vita trascorsi in cattive condizioni di salute sono dovuti a patologie associate ad obesità e sovrappeso. Cardiopatie ischemiche, ipertensione, *ictus*, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e carcinoma del colon sono tra le patologie in cui sono implicati il sovrappeso e l'obesità. Sovrappeso e obesità rappresentano per l'Europa una sfida sanitaria pubblica senza precedenti. Influiscono negativamente sulla salute psicosociale e sulla qualità della vita pubblica dell'individuo, ma rappresentano anche un costo rilevante per la sanità pubblica e, quindi, per la collettività. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'obesità negli adulti è responsabile in Europa cento della spesa in assistenza sanitaria. Le cause di tutto questo sono da ricercarsi nella generale modifica degli stili di vita alimentari; una tendenza crescente verso un consumo sempre maggiore di cibi a basso valore nutrizionale e, al contrario, ricchi di grassi e zuccheri, i cosiddetti cibi spazzatura o *junk food*, associati all'aumento del consumo di bevande zuccherate e ad una quotidianità sempre più sedentaria e scarsamente propensa all'attività sportiva. Dieta inadeguata e comportamento sedentario non devono essere considerati singolarmente, ma congiuntamente responsabili del carico sanitario. È, quindi, di fondamentale importanza che vi sia equilibrio tra un consumo misurato di cibi ad alto contenuto di grassi ed un'attività fisica costante. Indipendentemente dal peso, un'attività fisica regolare, anche moderata, influenza positivamente il metabolismo dei grassi e dei carboidrati e può ridurre notevolmente il rischio di diabete e della maggior parte delle altre malattie croniche più importanti. Secondo i dati dell'ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, la dieta inadeguata, la mancanza di attività fisica, la conseguente obesità e le malattie associate sono nel loro insieme responsabili di complicanze per la salute e mortalità precoce quanto il fumo di tabacco. Il sovrappeso incide dal 30 all'80 per cento negli adulti nella regione europea. L'aumento dell'obesità infantile è forse persino più allarmante. Oltre il 60 per cento dei bambini che sono in sovrappeso prima della pubertà lo saranno anche nella fase iniziale dell'età adulta. Questo riduce l'età media della comparsa di patologie non trasmissibili e influenza sensibilmente il carico dei servizi sanitari in quanto aumenta il numero di accessi e di prestazioni durante il periodo dell'età adulta. Il Ministero della salute ha attivato il sistema di sorveglianza OKkio alla Salute con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione dell'obesità infantile e valutare gli interventi di promozione della salute. L'analisi, relativa all'anno 2014, dimostra che il 20,9 per cento dei bambini italiani è in sovrappeso, mentre il 9,8 per cento è obeso, con una prevalenza più alta nelle Regioni del Sud e del Centro Italia. In particolare, l'osservazione delle abitudini alimentari associata all'analisi degli aspetti relativi al movimento e alla sedentarietà mostrano un quadro davvero poco incoraggiante. Uno degli aspetti sottolineati dallo studio riguarda la percezione che i genitori hanno degli stili di vita dei propri figli: poco più del 38 per cento dei genitori riconosce il grave sovrappeso e l'obesità dei propri figli e solo il 40 per cento ritiene che questi svolgano poca attività fisica. Numerosi studi hanno osservato un aumento di prevalenza di sovrappeso e obesità tra specifici gruppi di popolazioni identificati in base al livello di reddito o titolo di studio. Nella maggior parte dei Paesi della regione europea l'obesità è più frequente tra le comunità socialmente svantaggiate, caratterizzate da livelli inferiori di reddito, educazione e accesso all'assistenza.

e la percentuale destinata all'acquisto di alimenti è in calo. L'industria e i distributori di alimenti influenzano il consumo alimentare attraverso l'aspetto estetico, le dimensioni delle porzioni, la promozione di offerte speciali. l'Oms ha classificato come probabile, o comunque convincente, l'effetto negativo del *marketing* aggressivo dei cibi ad alta densità energetica sullo stato nutrizionale dei bambini e, anche se è necessario porre la massima attenzione al *marketing* rivolto ai minori, non si può sottovalutare la diversa capacità degli adulti di adottare scelte alimentari sane o di resistere ai richiami del *marketing*;

a prevedere un piano sanitario nazionale per una corretta alimentazione e, soprattutto, a stimolare un corretto stile di vita aumentando l'attività fisica.

L'obesità non è un fatto estetico, non può esserci un fai da te per contrastare l'obesità. l'obesità. Un obeso rischia di avere il 25 per cento in meno di aspettativa di vita, con patologie croniche invalidanti gravissime, diabete, malattie coronariche e percentuali consistenti di cancro. La vita dell'uomo, afferma il presidente dell'Istituto superiore di sanità, è inversamente proporzionale alla larghezza della sua cintura. Ciò è assolutamente vero. una pandemia molto preoccupante. Questa è una malattia complessa, cronica, invalidante, che ha bisogno di un approccio multidisciplinare. È una malattia con tanti fattori: è una malattia culturale e sociale, ma anche con aspetti genetici.

La dimensione del problema è talmente vasta e importante, che ha bisogno di tutta la nostra attenzione.

chiediamo che nel patto nazionale della prevenzione e il contrasto all'obesità 2014-2018

sono sottesi fenomeni economici particolarmente importanti, su cui invito ad una riflessione molto approfondita. L'obesità è una condizione medica, secondo me, e quindi non è una malattia,

ovviamente nella mozione n. 642 rimarchiamo che l'obesità rappresenta un problema patologico per un'alta percentuale della popolazione italiana che supera il 10 per cento. Si parla di una nuova cultura della scienza dell'alimentazione, di grasso tossico, di obesità come malattia cronica che porta a una riduzione degli anni di vita e ad un aumento esponenziale della spesa sanitaria. Si pensa che entro il 2030 in Italia gli il doppio di quelli che ci sono attualmente, il che porterebbe a triplicare la spesa per il Servizio sanitario nazionale e ciò significherebbe la insostenibilità.

di questo tipo di malattie che stanno imperversando nei pazienti delle strutture di riposo in Italia, con grande spesa sia familiare che del sistema sanitario nazionale. Quindi, il tema assume un'importanza ancora maggiore, alla luce soprattutto del *trend* crescente ed esponenziale che l'obesità fa I risvolti determinati da tale patologia solo in un primo momento sono di natura squisitamente medica. Altri colleghi hanno accennato alla necessità che il medico di base si impegni

intervento sarà contenuto anche perché chi mi ha preceduto ha illustrato in modo esaustivo le condizioni e le motivazioni

che naturalmente devono essere, sotto il profilo epidemiologico, valutati anche per area geografica. E così si scopre che l'incidenza dell'obesità e del sovrappeso si alza in termini percentuali nelle zone del Mezzogiorno d'Italia. Le implicazioni sono più devastanti della patologia stessa. Il paziente obeso va incontro a patologia diabetica, a cardiopatie ischemiche, ad arteriopatia e contrae più facilmente forme neoplastiche. L'obesità, ma anche il sovrappeso, incidono sulla qualità della vita e anche sulla quantità di vita. L'essere obeso clinicamente equivale ad uno stato di invecchiamento e l'OMS ci ricorda che la condizione di obesità riduce le aspettative di vita dall'8 al 15 per cento. I costi sono un aspetto si stimano complessivamente in circa 20 miliardi di euro nel nostro Paese. Naturalmente non ci sono solo i costi sanitari, ma ci sono anche quelli per la produttività persa, per il trasporto, per il capitale umano compromesso. Cosa chiediamo con la nostra mozione noi del Gruppo CoR? Chiediamo di attuare quegli interventi che nel nostro Paese sono stati ben definiti nell'ambito dei programmi di promozione della salute. Parlo dei piani nazionale e regionale di prevenzione, parlo del progetto Guadagnare salute o dello stesso Piano sanitario nazionale sulla malattia diabetica, che fa esplicito riferimento alla condizione dell'obesità. Il secondo punto è la necessità di attivare in modo continuativo e adeguato forme di sorveglianza e monitoraggio, che servono ad avere aggiornati i dati epidemiologici, anche al fine di una più corretta e puntuale misurazione degli effetti delle iniziative intraprese. Per questo potrebbe essere istituito un apposito gruppo di lavoro di alto valore scientifico. C'è inoltre la necessità di realizzare iniziative di informazione e di educazione. Il problema dell'obesità è senz'altro di natura di natura clinica, che ha primarie implicazioni di natura sanitaria, ma che affonda le sue radici primariamente in motivazioni che sono di tipo culturale e sociale. C'è poi la possibilità di valutare l'utilizzo *off label* del liraglutide, sulla cui efficacia terapeutica la comunità scientifica si è puntualmente espressa, e la necessità di incrementare il numero dei programmi volti a identificare i soggetti in condizione di obesità o di sovrappeso, promuovendo anche

Ritengo sia un bene che oggi l'argomento dell'obesità abbia avuto l'opportunità di essere discusso in quest'Assemblea, così da render nota la portata della questione e prospettare azioni di contrasto. È chiaro che tali questioni rappresentano un naturale problema di salute pubblica, di cui va evidenziata l'incidenza sulla spesa per il Servizio sanitario nazionale. Il mio intervento è incentrato soprattutto su due aspetti: quello della prevenzione e quello della riduzione delle disuguaglianze socio-economiche, perché in esse aumenta il livello di obesità e di sovrappeso. Comincio con il ricordare - come ha detto poc'anzi il collega che mi ha appena preceduta - che un bambino obeso sarà un adulto obeso, con il fondato rischio di comparsa delle malattie metaboliche che sono state più volte citate in quest'Assemblea. Quindi, il nodo centrale è la prevenzione, che svolge un ruolo importante: gli interventi precoci vanno promossi sin dal periodo del preconcepimento.

Dobbiamo considerare che noi viviamo in un ambiente che è veramente obesogenico e questo fenomeno è legato a più fattori citati anche in questa sede. Li ricordo solo per titoli: le abitudini alimentari scorrette e la diffusione di comportamenti sedentari.

sono praticamente inesistenti gli spazi pedonali grazie ai quali bambini e ragazzi potrebbero andare più facilmente a scuola a piedi, evitando di essere accompagnati ogni giorno dai genitori. O, ancora, alle attività ludiche, che tengono incollati i nostri bambini davanti al televisore o ai videogiochi: anche questo interferisce e determina il sovrappeso e l'obesità.

onorevoli colleghi, come ricordato nelle mozioni, le famiglie con meno cultura e meno abbienti tendono a mangiare di più cibi ricchi di grassi e carboidrati tralasciando più facilmente la cura del corpo, a partire dalla bocca. A causa di cibi con alto contenuto di zuccheri si abbassa il PH della bocca e i denti, se non vengono ben detersi e spazzolati dopo ogni pasto, si cariano. Sempre per mancanza di cultura e soldi, la bocca viene trascurata, con conseguente perdita di denti, i quali risultano essere utili per sorridere, per parlare e, ovviamente, per mangiare. La mancata triturazione del cibo, a causa di mancanza di denti, fa sì che le persone siano più propense a ingerire cibi più facilmente deglutibili, anche senza doverli masticare, e questi si riconducono a categorie di cibi ipercalorici e iperlipidici, quindi dannosi per l'organismo; combinati con la mancata triturazione, si ha un assorbimento maggiore del cibo a causa di una cattiva e rallentata digestione. Gli stessi fattori favorenti - cioè poca cultura e poca disponibilità economica

Lo sport aumenta l'azione della metmorfina, che serve a tenere bassa la glicemia, aumenta il colesterolo buono (HDL), che fa da spazzino e tiene pulite le arterie prevenendo l'ateromatosi e l'aterosclerosi vascolare; fa bene inoltre alla muscolatura e alle ossa, aiutandoci a mantenere più integro ed elastico il nostro scheletro e le nostre articolazioni. Io credo che per arrivare ad incentivare una corretta alimentazione e un corretto stile di vita, al fine di rendere il nostro Sistema sanitario nazionale sostenibile e, parallelamente, preservare la vita sana delle persone occorra agevolare la fruizione di cure e servizi, quali le cure odontoiatriche e la fruizione di palestre. Il modo in cui farlo sarebbe renderli accessibili economicamente attraverso un'offerta pubblica che copra la domanda. Lo si può fare, ma i tempi sono sicuramente troppo lunghi e onerosi. Partendo da ciò che già abbiamo, possiamo incentivare le cure e l'attività fisica attraverso le detrazioni delle spese. stabilità potrebbe essere fatta la scelta di favorire le cure odontoiatriche, dando la possibilità di detrarre il 53 per cento della spesa sostenuta e per chi fa attività sportive in palestre pubbliche o private o in associazioni

la possibilità di detrarre le spese per l'attività sportiva, in quanto la persona che la pratica ha meno rischi e necessità di ricorrere al Sistema sanitario nazionale

Il grasso corporeo si accumula quando il contenuto energetico di bevande ed alimenti supera l'energia richiesta dal metabolismo e dunque l'apporto energico ed il suo dispendio contribuiscono all'aumento del peso corporeo. quindi di fondamentale importanza che vi sia equilibrio tra un consumo misurato di cibi ad alto contenuto di grassi ed un'attività fisica costante. Indipendentemente dal peso, un'attività fisica regolare, anche moderata, influenza positivamente il metabolismo dei grassi e dei carboidrati e può ridurre notevolmente il rischio di diabete e della maggior parte delle altre malattie croniche più più importanti, con conseguente migliore qualità di vita e minori costi sanitari. È vero che non possiamo mangiare una vita da malati, come si dice a Firenze, per morire sani,

Presidente, è chiaro che i tempi particolarmente contenuti ci impongono di lavorare per *flash* e magari non si riesce a fare un discorso organico, però tutte tutte le mozioni che sono state presentate si sono rivelate puntuali nel trattare un argomento così importante e così scabroso. le cause che inducono l'obesità sono molteplici. Io le citerò *en passant* per poterci consentire, alla fine del nostro ragionamento, di fare alcune puntualizzazioni e richieste d'intervento parlamentari, ministeriali e governative che riteniamo importanti. Proprio in virtù di ciò che è stato già sottolineato - la scorretta alimentazione, la scarsa attività fisica, l'eccessiva meccanizzazione, la grande disponibilità di cibo, il progressivo aumento delle razioni, la diffusione di *videogame* e *social network*, la suscettibilità genetica,

si prevede un incremento significativo, in pochi anni, di obesi nella popolazione adulta. Vedete, si tratta di una malattia sociale in quanto determina isolamento di chi ne è affetto. Inoltre si associa ad importanti conseguenze sulla salute perché gli obesi sono esposti

o in sovrappeso, mentre la percentuale sale a circa il 34 per cento quando sono obesi o in sovrappeso entrambi i genitori. Dunque: l'obesità rappresenta un problema sociale ed economico che necessita l'intervento del Governo e del Parlamento.

si sta studiando un protocollo che riguarda la scienza dell'alimentazione. Vorrei sottolineare la bontà di tale intervento che deve essere consegnato alla Conferenza Stato-Regioni proprio per garantire

dipartimentale della prevenzione che aveva caratterizzato la presenza della medicina scolastica e dell'educazione sanitaria nelle vecchie USL. Abbandonando questo progetto organizzativo, purtroppo, si è rilevato un aumento abnorme

in due minuti non posso far altro che leggere che cosa ci raccomanda l'Organizzazione mondiale della sanità con le parole del suo direttore generale, Margareth Chan. Siccome

La sanità (...) deve fare i conti con l'industria del cibo (Big Food), delle bevande gassate (Big Soda) e alcoliche (Big Alcohol). (...) Pochi Governi danno la priorità alla salute rispetto ai grandi affari. Questo non è il fallimento della volontà individuale. È il fallimento della volontà politica di prevalere sul grande *business*». Credo che questo aspetto non sia stato ancora preso in considerazione.

raccomandare maggiore attenzione. Ricordo anche che è uscita da poco una revisione sistematica della letteratura sul trattamento farmacologico. Non vorrei che ci fosse anche Big Pharma che contrasta la possibilità di fare una battaglia contro l'obesità, perché i farmaci sono una dei tanti strumenti che

i nostri pareri saranno sostanzialmente in linea con quanto sto per affermare. Negli anni precedenti vi sono stati programmi molto importanti che sono stati anche citati, come Guadagnare salute

che tali condizioni fisiche possono determinare. Segnalo altresì che il Piano nazionale di prevenzione 2014-2016, nelle relazioni molto più stringenti che sono state costruite con le Regioni, prevede l'obbligo di compilare i piani regionali di prevenzione con un comitato di monitoraggio sul fronte degli obiettivi che si devono determinare.

una riformulazione del primo impegno: chiediamo che dopo la parola «sociali» venga aggiunta la dizione «limitatamente ai casi in cui l'obesità sia correlata ad altre patologie severe»,

chiediamo che venga aggiunta la formula: «a valutare la possibilità di». I punti 2) e 3) non sono condivisi dal Governo perché, come sarà sicuramente noto al senatore Gaetti, prevedono meccanismi di concertazione e di convenzione con i pediatri e che sono sottoposti a una formula di discussione e di dibattito democratico dal basso che noi possiamo sicuramente accompagnare, ma che non possiamo prendere in assoluta ed esclusiva responsabilità come Governo.

Signor Presidente, credo che il dibattito sia stato esaustivo, sia pure nei tempi contenuti. Le illustrazioni hanno toccato anch'esse in modo molto sintetico, ma efficace, le principali criticità; sono discretamente convincenti anche le repliche del Governo. Credo che su questa materia vadano mantenuti accesi i riflettori. Credo che il progresso della scienza non possa essere sottoposto al cono d'ombra di chi allunga sospetti anche sulla nostra Agenzia del farmaco, che ci fa fare bella figura nel mondo. che si prosegua con l'attività di ricerca di nuovi presidi terapeutici, senza dimenticare che la battaglia su questo versante si combatte sul fronte culturale culturale attraverso l'educazione, la sensibilizzazione e l'introduzione di efficaci campagne promozionali sui corretti stili di vita. a parlare il senatore Barani.

ancorché multidisciplinare, riteniamo sia d'interesse dello Stato e della salute dei cittadini che si ponga rimedio anche ai punti sollevati

a parlare il senatore De

introdurre una specifica imposta sui prodotti alimentari ad alto contenuto di grassi e basso valore nutrizionale e sulle bevande ricche di zucchero e anidride carbonica. So che

porterebbe a una diminuzione di 180.000 unità di cittadini britannici obesi e a un introito per le casse del Servizio sanitario britannico di 320 milioni di euro. Non voglio mettere in crisi l'economia di alcune aziende, ma sarebbe utile pensare

tre imprese su dieci hanno riformulato i propri prodotti rimuovendo completamente gli ingredienti critici, il 7 per cento delle imprese ha ridotto i livelli di zucchero, sale e caffeina una diminuzione del 27 per cento della vendita dei prodotti oggetto della tassazione che così costano di più (la gente che ha poche possibilità di spendere compra con più facilità il cibo spazzatura). Quindi, c'è stata una diminuzione del 35 per cento del loro consumo. Ringrazio, comunque, il Sottosegretario, e spero che nella giusta sede egli sia in grado di spingere il Governo verso questa visione della prevenzione e di far capire che il problema non si risolve pezzettino per pezzettino, ma in maniera globale.

Signor Presidente, anch'io ringrazio il Governo perché ha valutato attentamente le mozioni. Per quanto mi riguarda,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che l'obesità e tutte le patologie ad essa correlate siano diventate un problema serio su cui è necessario riflettere ed agire perché, come sottolineato nella mozione della collega Bianconi da me firmata, ha dei costi sociali ed economici sempre più alti ed è ormai un problema di prevenzione e sanità pubblica. Non voglio ripetere le cifre impressionanti già illustrate, ma le campagne di informazione e di contrasto che si sono via via succedute in diverse Nazioni fanno capire quanto sia necessario prestare la massima attenzione a quella che potremmo definire come una «sindrome da società del benessere». Anche se è vero che non solo nei Paesi «ricchi» si sta alzando la percentuale di obesità, certamente una migliore possibilità di accesso al cibo e la scarsa propensione alla mobilità fisica incrementano in maniera esponenziale il rischio di eccesso di grasso corporeo. l'obesità è un fattore di rischio per tutte le malattie ad essa correlate: in particolare, mi riferisco al diabete e alle malattie cardiovascolari. In Europa dagli anni Ottanta è triplicato il numero di bambini obesi, soprattutto in Italia, che vanta il triste primato del secondo posto al mondo.

su 830 bambini ha fatto osservare come l'incremento del grasso corporeo a otto e dieci anni predice sensibilità all'insulina nei due anni successivi. L'incremento del tempo trascorso davanti allo schermo peggiora la dinamica dell'insulina. Quindi, certamente è il momento di agire. Le nostre mozioni sollecitano il Governo in questo senso. Non siamo d'accordo sulla tassazione del cosiddetto cibo spazzatura e delle bevande zuccherate, anche perché abbiamo l'esempio del Regno Unito, dove ci sono i bollini rossi su prodotti italiani, come può essere l'olio d'oliva. Pertanto si tratterebbe di penalizzare un settore e favorirne un altro e questo non influirebbe minimamente sulla salute. Le cose importanti sarebbero l'informazione e il controllo. Credo infatti che il Ministero della salute dovrebbe intraprendere un'azione seria con il MIUR affinché ci sia un controllo sulle mense scolastiche. È inaccettabile vedere come in alcuni asili

vigilare, oppure fare educazione e lasciare distributori di merendine e bibite alla portata di tutti. Avete ascoltato le cifre del costo economico per il nostro Paese; è una situazione sicuramente molto grave.

Si deve cercare di indicare nell'associazione di dieta e attività motoria la migliore risposta all'obesità. Quindi, devono

Nella mia dichiarazione di voto vorrei sottolineare brevemente alcuni aspetti che sono stati presi in esame nel dibattito, ma su cui penso sia molto importante ritornare. Siamo tutti d'accordo che la battaglia contro l'obesità sia diventata prioritaria; essa vede l'impegno

un punto di riferimento importante nella necessità di intraprendere percorsi sostenuti che riguardino la modificazione degli stili di vita e una giusta alimentazione.

C'è un aspetto che vorrei sottolineare, concordando sull'idea che la prevenzione sia l'elemento fondamentale e che non dobbiamo rischiare di affrontare il tema dell'obesità sotto il profilo della medicalizzazione perché poi questo, come sottolineava la senatrice Dirindin, rischia anche di favorire e agevolare nell'immaginario collettivo l'idea che ci si possa

alimentare. Ciò aiuta a combattere il fenomeno, sempre più diffuso nel nostro Paese, che è quello del rifiuto del proprio corpo, con l'attribuzione all'immagine fisica, alla presentazione fisica del corpo degli adolescenti, un significato che non

per parti separate.

Signor Presidente, informo gli onorevoli senatori che ho appena depositato l'intervento stenografico che il Presidente del Consiglio ha tenuto alla Camera dei deputati. Credo tuttavia che possa essere utile aggiungere alcuni elementi informativi specifici legati

Ricorderò anche alcuni punti chiave dell'intervento del Presidente del Consiglio e quindi del Governo. Il primo certamente è il nostro impegno a far uscire l'Unione europea dall'attuale frenetico immobilismo, cioè da uno *status quo* che non permette di alzare il ritmo e di alzare le ambizioni politiche dell'Unione europea, come invece il Governo italiano intende fare. È questo il vero motivo della nostra valutazione negativa del vertice di Bratislava, in cui non è accaduto niente di significativo, come ha detto per primo il Presidente del Consiglio, subito dopo quel vertice informale. Una settimana dopo, praticamente con le stesse parole, lo ha confermato in sede istituzionale europea il presidente della Commissione europea Jean-Claude Junker. Quindi, per quanto riguarda quel processo che doveva partire a Bratislava, che si snoderà attraverso i due Consigli europei (il primo è quello di cui parliamo oggi, mentre il secondo è previsto a dicembre) e che troverà un momento importante, almeno nelle ambizioni e nelle intenzioni del Governo italiano, a Roma nel 2017 (quando, il 25 marzo del prossimo anno celebreremo i sessant'anni del Trattato di Roma), diventa ancora più importante alzare il ritmo e il livello delle ambizioni politiche.

ha annunciato avverrà nel marzo 2017. Non possiamo stare fermi in attesa dell'articolo 50, ma dobbiamo lavorare a 27 per fare veramente di Roma 2017 un successo, per tenere alte le ambizioni che noi abbiamo per Roma 2017, che consideriamo un momento fondamentale. Lo consideriamo fondamentale soprattutto pensando ai giovani europei e anche ai giovani britannici con riferimento alla Brexit, i giovani che erano andati a votare avevano votato massicciamente a favore del *remain*, ossia della decisione del Regno Unito di rimanere nell'Unione europea. L'altro aspetto molto rilevante è la volontà del Governo di lavorare insieme per preparare Roma 2017. Lavorare insieme significa lavorare con tutti i Gruppi politici ed è l'invito che a nome del Governo rivolgo al Senato, come il Presidente del Consiglio ha fatto alla Camera. Noi in Europa non rappresentiamo la maggioranza, ma rappresentiamo, con orgoglio, la Repubblica italiana e riteniamo che, quando in Europa stiamo preparando momenti importanti come il rilancio del processo di integrazione politica europea in occasione dei sessant'anni del Trattato di Roma, sia assolutamente auspicabile e opportuno - e questi sono gli auspici del Governo - lavorare insieme ai Gruppi politici di maggioranza e di opposizione

a Roma 2017, di avviare un dialogo forte e di coinvolgere quei deputati europei che sono stati e sono relatori di importanti rapporti parlamentari che riguardano il futuro dell'Unione europea e le modalità con cui rilanciare il processo di integrazione politica. Mi riferisco al rapporto degli onorevoli Bresso e Brok su come rafforzare l'integrazione politica sfruttando pienamente i trattati esistenti, ai rapporti Berès e Böge su come rafforzare una *governance* economica, sociale e democratica, soprattutto nella zona euro, e al rapporto Verhofstadt sul futuro dell'Unione europea. Vogliamo, quindi, avviare un rapporto molto forte di cooperazione anche con il Parlamento europeo

legato al futuro dell'Unione europea: è il processo di revisione del quadro finanziario multiannuale, cioè, in parole più comprensibili, il processo di revisione del bilancio europeo. In questo momento stiamo riesaminando il quadro finanziario da qui al 2019, ma all'inizio del prossimo anno si avvierà il processo per rivedere in maniera più ampia il bilancio dell'Unione europea nel periodo che andrà dal 2019 in poi.

di quei Paesi che oggi invocano la solidarietà quando si tratta di politiche di sviluppo regionale e di ricevere ingenti mezzi finanziari dal bilancio dell'Unione europea per il loro sviluppo regionale, che poi dimenticano improvvisamente il valore politico e giuridico della solidarietà quando si tratta di rispettare i diritti fondamentali e, in particolare, gli impegni assunti a livello europeo in materia di immigrazione e di diritto d'asilo. Riteniamo - ed è stato detto anche nelle sedi europee più formali - che il principio di solidarietà flessibile sia una contraddizione in termini. Conosciamo, come ho detto, il principio di solidarietà; conosciamo - e lo conosce anche questo Parlamento - il principio di flessibilità, sia per quanto riguarda il Patto di stabilità e crescita, sia per quanto riguarda il funzionamento del bilancio europeo, ma il principio di solidarietà flessibile, che da alcuni Paesi è stato proposto a livello europeo, non appartiene né agli impegni giuridici e ai trattati europei, né a politiche europee che noi possiamo condividere.

e che elaboreremo insieme, anche con il contributo del Parlamento italiano, e che vorremmo far valere nel momento in cui avvieremo la revisione del bilancio dell'Unione europea. Questi, Presidente, sono i punti chiave dell'intervento del del Presidente del Consiglio, che ha voluto ricordare in chiave di politica internazionale e di alto momento di politica estera, la sua visita a Washington, che avverrà da lunedì a mercoledì prossimo e, citando le parole di Obama, ha ricordato che nella valutazione del Presidente degli Stati Uniti, il rapporto Italia-USA raggiunge oggi il livello più alto della sua storia. Credo che di questo dobbiamo essere certamente tutti orgogliosi, come Italia, vista l'importanza che, ne sono sicuro, tutti i Gruppi politici attribuiscono al rapporto politico e alla forte alleanza che ci lega da settant'anni con gli Stati Uniti. Signor Presidente, prima di terminare vorrei aggiungere alcuni aspetti che sono relativi,

Questo Consiglio europeo si concentrerà su alcuni grandi aspetti e il primo certamente sarà quello dell'immigrazione. Sembra che, rispetto a Bratislava, nelle intenzioni ci sia un po' più di coraggio, quantomeno si dà maggiore importanza all'Africa. Si indica esplicitamente l'importanza di sviluppare un nuovo partenariato nelle immigrazioni tra Europa e Africa. All'interno di tale partenariato, che deve essere ampio e deve basarsi su nuove politiche di sviluppo attraverso investimenti pubblici e privati in cambio di un impegno maggiore da parte dei Paesi di origine e di transito sull'immigrazione, c'è ovviamente anche il tema dei rimpatri, che noi vogliamo collegare ad un risultato importante per l'Italia e cioè l'inizio di attività, entrata in vigore Guardia costiera e di frontiera europea. È un'iniziativa che noi, lo ricorderete, avevamo preso durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. Avevamo indicato allora, devo dire nello scetticismo generale a livello europeo, la necessità di creare una forma di integrazione molto più forte tra le posizioni di frontiera per cominciare a gestire in maniera più efficace le frontiere esterne; oggi questo è una realtà e noi vogliamo che diventi immediatamente operativa e funzionale in tutte le frontiere esterne, a partire dal Mediterraneo. Si discuterà al Consiglio europeo anche del piano di investimenti esterno, quello che è stato definito il piano Juncker per l'Africa, vale a quei fondi e quel sistema di garanzia aggiuntivo che devono essere lo strumento finanziario della nostra strategia del *migration compact*, cioè di un nuovo partenariato per l'immigrazione e lo sviluppo tra Europa e Africa. all'interno dell'immigrazione, faremo valere la nostra insoddisfazione, più volte manifestata dal Governo, per la mancanza del rispetto delle decisioni sulla redistribuzione dei richiedenti asilo ancora molto insufficiente quello che sta accadendo in Europa), così come insisteremo perché si prosegua, con ancora maggiore intensità,

non devo ricordarlo - è uno dei pilastri della strategia nostra ma anche di quella che dovrebbe essere la nuova strategia europea in materia di immigrazione e di asilo. L'altro aspetto è quello relativo al commercio. Si valuterà

erano state rivolte al Governo, c'era proprio quello di assicurare una centralità dei Parlamenti nazionali su questo. Discuteremo anche dell'introduzione di nuovi strumenti di difesa commerciale delle imprese europee - e quindi delle imprese italiane - a livello globale. Riteniamo che rafforzare gli strumenti di difesa commerciale non sia neoprotezionismo, ma significhi dotarci di strumenti

compiendo. Questo non ci impedirà di continuare a seguire e fornire orientamenti strategici sulle singole proposte legislative, che sono di grande rilevanza per l'Italia. Penso ad esempio al *dossier* sull'Effort sharing. Il tema della crescita e del mercato unico sarà uno degli argomenti fondamentali su cui si dovrà fare una valutazione

è importante che, entro la fine dell'anno, si prenda la decisione formale di raddoppiare il piano di investimenti strategici, il cosiddetto Piano Juncker, rispettando l'impegno che il Presidente della Commissione europea ha preso davanti al Parlamento e che noi con forza sosteniamo. *(Applausi

Nel frattempo, però, in quest'Aula si è votato. Se non erro, noi senatori siamo ancora legittimati ad esprimere un voto,

Questa è la situazione e non è oggetto di discussione: c'è una decisione già presa dalla Conferenza dei Capigruppo, comunicata all'Assemblea e su cui si è votato. Su questa votazione nessuno ha obiettato alcunché

forse i Presidenti di Commissione, a questo punto, dovrebbero essere un po' più accorti e concordare con la Presidenza gli orari in cui far venire i senatori in Aula a votare. Si trattava solamente di dieci minuti, non di più. Non ne faremo un caso nazionale: è una cosa che speriamo finisca

Signor Presidente, se lei trasferisce un piccolo incidente alla sensibilità della Presidenza della Commissione,

che il nostro Paese arrivi alla riunione del Consiglio europeo, purtroppo, profondamente sconfitto. Credo convenga evitare ipocrisie e dirlo con grande nettezza, apertamente, così come conviene dire molto onestamente che in questa sconfitta il nostro Governo ha purtroppo diverse responsabilità. Abbiamo chiesto più volte di rivedere quel Regolamento di Dublino che obbliga i migranti - il Sottosegretario ne ha fatto cenno - a essere registrati e a rimanere nel Paese di prima accoglienza e che, quindi - come sappiamo - penalizza l'Italia e la Grecia più di chiunque altro. Purtroppo, non siamo stati ascoltati e il nostro Governo non ha nemmeno replicato più di tanto. Avevamo parlato a lungo, anche in questa sede, di mettere in campo una strategia completamente differente, più umana, allo stesso tempo anche più efficace e giusta, che fosse basata - ad esempio - su corridoi umanitari e sul diritto di asilo, ma anche su questo siamo stati ben poco ascoltati, anche perché abbiamo fatto davvero molto poco per esserlo. Più che a garantire ai profughi un'accoglienza civile e a difendere i legittimi interessi dell'Italia, il nostro Governo è stato molto attento a disturbare molto poco il possibile manovratore. Del resto, forse non poteva fare diversamente, dal momento che, dietro le belle parole e anche qualche denuncia verbale, la sua strategia economica si basa sulla benevolenza di quei manovratori, sulla disponibilità cioè dell'Europa a chiudere un occhio, a volte addirittura entrambi gli occhi, sullo stato reale dei nostri conti. Noi purtroppo siamo di nuovo in una situazione drammatica, anche se probabilmente si fa finta di non vedere fino in fondo la Le previsioni contenute nel DEF sono state rivedute al ribasso e, anche così, per parere unanime, sono molto più rosee del dovuto. tra tutti i Paesi europei siamo probabilmente quello che trae meno vantaggi dalla piccola ripresa in atto. In appena sette mesi, il debito pubblico è cresciuto di oltre 80 miliardi di euro e questo è davvero un *record* assoluto. Anche il fallimento del *jobs act* è talmente evidente che persino una stampa molto compiacente, come quella che, purtroppo, spesso si occupa delle questioni politiche nel nostro Paese, deve prenderne atto. Per non parlare poi della disoccupazione giovanile, che resta a livelli altissimi e non è nemmeno scalfita da quegli incentivi pagati da tutti quanti noi alle aziende. Naturalmente, conosciamo la conseguenza, non è notizia di oggi e non abbiamo minimamente invertito la tendenza nemmeno negli ultimi mesi: mesi: diverse decine di migliaia di giovani (100.000 nell'ultimo anno) con livello di formazione alto, altissimo in qualche caso, abbandonano il nostro Paese. Per attrarre gli investimenti esteri il Governo può vantare un'unica cosa: mettere in campo un costo del lavoro più basso tra i Paesi in condizioni simili al nostro. Non ci vuole molto a capire che questa è davvero la via peggiore e, in prospettiva, più controproducente. Si tratta davvero di una sorta di indice di declino vicino alla irreversibilità. Questa situazione così drammatica non è soltanto responsabilità di una congiuntura internazionale peggiore del previsto, ma è anche frutto di una politica sbagliata,

e ora, che è imminente il *referendum* costituzionale, probabilmente la manovra servirà ancora una volta a distribuire qualche regalo, nella speranza di conquistare così il voto degli italiani. italiani. Un Governo che deve chiedere all'Europa di non vedere lo stato reale dei suoi conti e di perdonare i regali elettorali non può poi permettersi più di tanto di insistere affinché - per esempio - il Regolamento di Dublino venga seriamente modificato o perché l'emergenza profughi venga affrontata in modo strutturalmente diverso. Al massimo, il Governo può far finta di strillare, come ha fatto stamattina

e ritengo estremamente sbagliato che il commissario Moscovici abbia giustificato la sua posizione non con un ripensamento a proposito della sciagurata politica del rigore, che ha segnato drammaticamente la storia degli ultimi anni fino a produrre il disastro nel quale siamo sprofondati oggi, e neppure con i risultati ottenuti dall'Italia, ma con la necessità - udite bene - di sostenere il Governo italiano contro presunte forze populiste. Ecco: a me sembra davvero inaccettabile immaginare che si possa ammettere che la flessibilità vada concessa all'Italia non per risolvere le sue questioni strutturali, ma per aiutare il nostro Governo a vincere il *referendum.* Mi pare un'ingerenza insopportabile ai danni di una libera consultazione democratica

La politica del rigore si è dimostrata disastrosa in tutti questi anni e per questa ragione, deve essere abbandonata. Usare la concessione della flessibilità per avvantaggiare una parte politica piuttosto che l'altra, un fronte referendario piuttosto che l'altro, costituisce un'intromissione che in un Paese libero tutti dovremmo essere in grado di

in cui i cittadini di questo Paese devono potersi esprimere non su questioni di contorno, ma su elementi decisivi che riguardano la vita politica nazionale. Signor Presidente, per l'ennesima volta in quest'Aula il Presidente del Consiglio rinuncia ad essere presente e implicitamente rinuncia al suo ruolo per portare avanti una deleteria campagna referendaria per il sì, quando il Paese è nel pieno di un'emergenza economica. L'esigenza del *Premier* di dover necessariamente cambiare la Costituzione è l'esempio della distanza siderale della vostra politica dai bisogni del Paese. È per questo che perderete il *referendum* e andrete a casa. Ritorniamo al tema di oggi: come dicevo, per l'ennesima volta in quest'Aula si parla di migranti, di trattati commerciali internazionali e di rapporti con la Russia. Per l'ennesima volta, in quest'Aula si ripropongono le stesse ricette, che hanno dimostrato di essere fallimentari e di produrre danni al Paese. È il caso della politica estera dell'Unione europea, che di fatto produce una mole impressionante di profughi, aumentando in maniera ingiustificata le tensioni con la Russia. Oggi parliamo di emergenza migranti perché nel 2011 il PD, partito che sostiene questo Governo, ha premuto per bombardare la Libia di Gheddafi, creando il caos. Oggi, signor Sottosegretario, siamo ostaggio delle milizie islamiche di Misurata, siamo costretti a supportare un *Premier*, al-Sarraj, che in Libia non è riconosciuto da nessuno ed è costretto a nascondersi in una base navale a Tripoli, in pieno contrasto con la risoluzione ONU, che - voglio ricordarlo - non diceva di formare un Governo a tutti i costi, di innestare un *Premier* fasullo in un Paese in guerra, ma aveva stabilito una *road map* che vedeva un accordo tra il Governo di Tobruk e quello di Tripoli, cosa che non si è mai verificata. Così, pian piano, da *Premier* designato, al-Sarraj è diventato semplicemente *Premier* e oggi la Libia è ripiombata nello stesso caos del 2014, mentre il povero ministro Gentiloni è costretto a correre a destra e a manca per supportare un Governo fantoccio calato dall'alto e sabotato da egiziani, francesi, inglesi e turchi. Questo è lo stato dell'arte. In questa situazione vorreste addestrare la Guardia costiera libica; ci vuole qualcuno che vi ricordi che della Guardia costiera libica non vi è neanche l'ombra. Piuttosto state addestrando la marina delle milizie islamiche di Misurata, su cui pendono pesanti sospetti nella gestione del traffico di esseri umani. Signor Signor Presidente, che paradosso: finanziamo quelli che potrebbero essere i trafficanti di esseri umani che tanto vogliamo combattere. Verrebbe da ridere se in mezzo non ci fossero le vite di migliaia di persone che arrivano in Libia dall'Africa e che da quella Libia, in cui prima del 2011 si fermavano a lavorare, ora scappano a gambe levate per evitare di finire nelle mani delle milizie che voi, insieme ai vostri alleati/nemici inglesi, francesi, egiziani, turchi e sauditi, state finanziando. La stessa cosa possiamo dire sulla Siria, Paese pacifico che fino al 2011 non aveva un solo profugo e che, grazie alla vostra insopportabile retorica umanitaria, ai finanziamenti e alle armi che avete concesso con il gruppo "Amici della Siria", ora è devastata da quasi sei anni di guerra. Nel 2011 dalla Siria non usciva un profugo, oggi in giro ce ne sono quasi 4 milioni, più altri 6 dentro il Paese. Non parliamo dell'Africa, da cui arrivano centinaia di migliaia di persone grazie all'operosa azione delle nostre multinazionali, intente a finanziare regimi sanguinari e a spolpare le risorse del Continente. Quelli che voi chiamate migranti economici sono in qualche modo profughi di una guerra coloniale a bassa intensità, che depreda risorse dai tempi delle opere di civilizzazione coloniale in maniera ininterrotta. Eccoci al dunque: come possiamo affrontare il tema dei migranti senza affrontare la politica estera dell'Italia e dell'Unione europea? Partiamo dunque dalla politica estera e, per essere meno vaghi, partiamo dalle sanzioni alla Russia. Il Movimento 5 Stelle non ha mai sostenuto le sanzioni alla Russia perché vediamo questo Paese come un alleato in almeno due campi. Sul campo economico, l'Italia aveva un significativo *export* verso la Russia. Con le sanzioni abbiamo perso, secondo le stime, circa 1,5 miliardi; un un autogol clamoroso, che tra l'altro non ci ha portato alcun beneficio in termini geopolitici. Abbiamo isolato infatti i russi per accogliere un Governo nazifascista ucraino che perseguita i propri cittadini di origine russofona e apporta zero euro alle nostre casse. L'altro aspetto che riguarda i rapporti con la Russia è legato alla lotta al terrorismo. Infine i russi, in un anno, hanno fatto più di quanto abbia fatto la "coalizione dei volenterosi" in cinque. L'ISIS, creatura oscena, finanziata dai sauditi, armata e addestrata da mezzo mondo occidentale, ha perso 586 villaggi e città e 12.360 chilometri Oggi il sogno di un califfato islamico non è più realizzabile grazie ai russi, non certo ai *raid* della coalizione. Noi del Movimento 5 Stelle chiediamo allora di togliere le sanzioni alla Russia e di formare una coalizione internazionale contro il terrorismo che comprenda anche i russi. Democratico, ci sta o no? Nello stesso tempo, chiediamo al Governo di agire sull'immigrazione irregolare in due direzioni: per quanto riguarda la Libia di ascoltare i sindaci libici, che mi creda, signor Presidente, in quel Paese martoriato sono gli unici a essere passati dalle elezioni. Presidente, per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti chiediamo di spingere l'Europa a cambiare rotta: che senso ha mantenere una flotta militare, quando l'emergenza è soccorre i migranti? Abbiamo visto foto di migranti stipati a poppa delle navi militari, stretti gli uni con gli altri. Le navi militari sono fatte per combattere, e non per salvare i migranti. Per questo chiediamo al Governo di spingere l'Europa affinché la missione navale militare sia trasformata in missione civile. Ci vogliono traghetti non navi militari per soccorrere i migranti. Su questo punto il Movimento 5 Stelle è disposto a discutere forme e modalità, a patto che le finalità siano il risparmio, il soccorso in mare efficace e una diversa politica di redistribuzione degli arrivi. Il terzo punto è l'accoglienza. Avete creato un sistema confuso e inumano sia per i migranti che per i cittadini italiani, da un giorno all'altro si vedono calare dall'altro strutture di accoglienza che costano un occhio della testa e creano ricchezza solo ai pochi che le gestiscono. Noi proponiamo di pagare delle somme in compensazione ai Comuni che accolgono i migranti, in ragione dei disagi sociali che la popolazione e il Comune che accoglie subiscono. Se un Comune accoglie i migranti, oltre alle spese di gestione, deve ricevere dei soldi da spendere in servizi sociali per i propri cittadini, deve essere esonerato dal rispetto del Patto di stabilità per quelle somme e deve poter portare dei benefici per il territorio. Allo stesso modo i servizi di assistenza ai migranti, l'alloggio, il cibo e quanto necessario devono essere forniti dalle piccole e medie imprese del territorio, non da cooperative che solo lucrano sui migranti. Vedrete come i Comuni e i cittadini saranno felici di accogliere i migranti a queste condizioni. Voi invece, con questo sistema, foraggiate il razzismo e la corruzione. Questi soldi li deve corrispondere l'Unione europea e non il Governo italiano e voi avete il dovere di andare in Europa e battere i pugni sul tavolo, senza pantomime alla Renzi, per capirci.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, gli argomenti che lei ha trattato a nome e per conto del Presidente del Consiglio

- il Presidente del Consiglio ne ha parlato alla Camera dei deputati e lei, signor Sottosegretario, anche per questioni di tempo, ci farà sapere nella replica - e lo stato dell'arte, che è ancora ai primi

particolarmente odiosa e che si scarica essenzialmente sui Paesi di frontiera, come Italia e Grecia, renda di fatto impraticabile ogni possibile soluzione. Quindi,

essere valutata in circa 6 miliardi di euro; la perdita di questo mercato ha riguardato gran parte del "*made in*" concentrandosi, particolarmente, sull'agro-alimentare, con una penalizzazione che ha riguardato l'intero Paese, ma prevalentemente il Mezzogiorno il tutto mentre la domanda estera, che nel 2012 e 2013 aveva esercitato un ruolo traente, che attenuava i morsi dell'*austerity*, a partire dal 2014 ha subito una netta inversione di tendenza, costringendo la politica economica italiana a far conto più sulla domanda interna che non sul sostegno delle esportazioni,

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, c'è un passaggio dell'intervento del presidente Renzi alla Camera dei deputati che mi ha particolarmente colpito, ossia l'attenzione che l'Europa deve avere per l'Africa e l'incredibile amnesia del documento di Bratislava. Alcune settimane fa, partecipando al vertice della sottocommissione NATO a Il Cairo, il rappresentante del Ministero degli esteri egiziano si è lamentato con noi per come l'Europa abbia sostanzialmente disatteso l'Accordo di Malta del novembre 2015, con cui ci si impegnava a fornire risorse e strumenti per il controllo dei flussi migratori e per lo sviluppo dei Paesi africani, in una cornice complessiva anche di gestione dell'emergenza umanitaria e dei profughi. Questo è solo un esempio, ma rende bene l'idea di un'Europa che troppo spesso - per usare le parole del Presidente del Consiglio - sembra mossa da un frenetico immobilismo; lo stesso che ritroviamo sui conti, sul riconoscimento di una certa dose di flessibilità economica per i Paesi come il nostro, che sono chiamati a gestire eventi straordinari e drammatici quali il terremoto, la gestione dei flussi migratori, ma anche la lotta al terrorismo. Gli egoismi nazionali e i veti non servono a niente e non sono giustificabili. Alcuni Paesi - e mi riferisco soprattutto a quelli dell'Est - che usufruiscono di fondi strutturali e vengono aiutati in settori come quello industriale e agricolo, non possono poi non dare la loro solidarietà quando l'Europa affronta una grave crisi migratoria. Per fortuna ogni tanto qualche luce c'è. solo citare due eventi recenti: il via libera dato da Strasburgo, senza aspettare l'approvazione formale dei singoli Governi, per l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi sul clima e per il contenimento del riscaldamento globale, ma anche l'iniziativa, estremamente meritoria, dell'Interrail gratuito per i diciottenni, un'occasione per conoscere, capire, aprire lo sguardo, per sentirsi tutti figli di un'unica casa europea. Tuttavia, ciò non basta: oggi l'Europa è attraversata da populismi che fanno tremare le gambe per la loro volontà di rialzare muri, che minerebbero - è proprio il caso di dirlo - le stesse fondamenta del sogno europeo. Brexit, Polonia, Austria, il *referendum* ungherese e le elezioni amministrative in Germania: l'elenco è molto lungo e speriamo davvero di non aggiungere anche il dibattito sul *referendum* costituzionale, con quella spirale perversa del tanto peggio, tanto meglio che purtroppo vedo aleggiare, quando invece si dovrebbe ragionare seriamente e serenamente nel merito della riforma e dell'occasione che essa può costituire per la semplificazione del sistema. che trova alimento nell'incapacità dell'Europa di essere stata un punto di riferimento soprattutto durante gli anni difficili della crisi e che non riesce a scrollarsi di dosso quest'immagine. Mi ha molto colpito scoprire che il Paese che, dopo un anno dall'entrata in vigore del piano Juncker, è riuscito a intercettare la quota più cospicua di risorse è stato proprio il Regno Unito, seguito a stretta distanza dall'Italia. È la riprova che - al di là degli aspetti economici che sono assolutamente importanti e su cui fa benissimo il nostro Governo a tenere il punto - l'Europa paga gravemente le divisioni tra i Paesi, l'assenza di una forte unità d'intenti per gestire situazioni gravi e complesse, come quelle che abbiamo enunciato. Per questo è assolutamente condivisibile la battaglia che questo Governo ha sempre fatto in sede europea per liberare le risorse destinate ad archiviare la stagione dell'austerità: le regole servono per raggiungere gli obiettivi e non viceversa. Purtroppo, anche la Provincia autonoma di Trento oggi si trova, per colpa di norme sbagliate, un avanzo di bilancio a rischio congelamento, laddove l'unica colpa è quella di aver saputo gestire con attenzione ed efficacia il proprio bilancio. Se ne parlerà in altra sede, ma anche questo è un punto molto importante su cui chiedo l'impegno del Governo a risolverlo. Trovo condivisibile l'atteggiamento complessivo dell'Esecutivo in Europa sui flussi migratori, sulla ricerca di una nuova autorevolezza. L'Europa deve arrestare la corsa alla demolizione, frutto degli egoismi nazionali, per tornare a essere il luogo della speranza, il punto di riferimento per le generazioni per le generazioni del futuro. L'Europa è la più grande intuizione politica del Novecento, ma oggi è soprattutto un attore necessario e indispensabile nella complessità di un mondo multipolare, attraversato da guerre tremende, un mondo che vede Paesi come la Cina entrare in una fase nuova, del tutto inedita sul piano economico e in parte sul piano sociale; un mondo che deve sapersi misurare e confrontare con la Russia di Putin.

purtroppo ci riporta a quanto sta accadendo in Europa. C'è un'ultima iniziativa che forse il presidente Obama può fare per il nostro Paese. Parlo di Chico Forti, un cittadino italiano con una vicenda giudiziaria ricca di elementi oscuri, su cui lo scorso anno la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità una mozione per la riapertura del processo. simile ho presentato io stesso qui in Senato ed è stata sottoscritta e condivisa da decine di colleghi; non sono inoltre mancati gli appelli al presidente Mattarella, affinché avviasse un'iniziativa diplomatica per chiedere la grazia. La vicenda di Forti continua a interessare e a scuotere una parte significativa della nostra opinione pubblica e in particolare quella del Trentino. Spero allora che il Presidente del Consiglio, anche sulla scorta della mozione votata alla Camera e del documento presentato in Senato, vorrà cogliere quest'occasione per sottoporre la questione al presidente Obama.

Governo, colleghi, siamo alla vigilia dell'ennesimo Consiglio europeo e dobbiamo ammettere che lo spirito è di crescente rassegnazione di fronte a un'Europa sempre più chiusa in se stessa e prigioniera delle paure dei singoli Paesi. Dopo la Brexit ci si poteva aspettare (anzi, ci si aspettava) una presa di coscienza e uno scatto in avanti verso una maggiore coesione. Anche l'incontro per ricordare Altiero Spinelli e il suo manifesto per un'Europa unita ci ha fatto sperare che tre grandi Nazioni come Francia, Germania e l'Italia avessero fatto tesoro della decisione del popolo inglese di uscire dall'Unione europea, decidendo finalmente di cambiare rotta, di intraprendere una linea politica differente oltre che più chiara e unitaria. nonostante gli sforzi del Presidente del Consiglio e del Governo, ciò non è avvenuto. Al contrario viene alla luce un vuoto di idee a causa della posizione difensiva di alcuni Paesi, soprattutto Francia e Germania, in attesa di imminenti elezioni, che mette davvero a rischio l'Unione europea e il suo futuro civile e democratico. è inutile negare che oggi l'Europa è solo un insieme di politiche nazionali, in alcuni casi persino di nazionalismi e di pericolosi sciovinismi. L'Italia in questo contesto è un modello virtuoso, anche se veniamo lasciati soli ad affrontare problemi giganteschi, sui quali, per di più, si avventano estremisti e populisti di casa senza scrupoli. Ritengo, infatti, un grave errore delle forze democratiche in Europa, impaurite dalla destra che avanza speculando sulle paure dei cittadini, rimandare decisioni importanti piuttosto che rilanciare subito, con determinazione, le idee che sono alla base dell'Europa unita e solidale. Il Presidente del Consiglio e il Governo hanno davanti un percorso davvero impervio; devono affrontare diverse difficili sfide - ma tutte legate fra loro - per il futuro del nostro Paese. la sfida dell'Europa, dove l'Italia ha certamente un ruolo fondamentale, ma non esclusivo, perché serve anche l'impegno e la determinazione delle forze democratiche degli altri Paesi europei e dei loro *leader*, che devono dimostrare di essere dei veri *leader* che non barattano i loro principi per la paura dell'avanzata dei populismi, e poi c'è la sfida interna dell'Italia: l'Italia che ha bisogno di un salto, di un cambiamento vero; l'Italia che ha bisogno di dimostrare a se stessa, prima ancora che al resto del mondo che è lì in attesa di vedere cosa accadrà il 4 dicembre, di saper voltare pagina e guardare al futuro. Anche questa sfida non dipende solo dalle forze politiche che sostengono la riforma e dal presidente Renzi, che si sta battendo per l'approvazione della riforma costituzionale con tutte le sue forze (e ciò gli fa onore perché si sta battendo non per una sua vittoria ma per una vittoria del Paese e di tutti gli italiani). Questo gli italiani lo devono sapere. Ecco perché dipende soprattutto da loro: è una battaglia che riguarda il loro futuro, non quello del Governo, e che devono vincere loro. loro. L'approvazione di questa riforma rappresenta un'occasione per svoltare davvero pagina, chiudendo il capitolo del passato e guardando al futuro con più maturità, forza e capacità di costruire un'Italia migliore all'interno di un'Europa migliore. PRESIDENTE.

infatti che sia eccessiva la rilassatezza, se non la rassegnazione, con la quale si vivono novità rilevanti come quella di prevedere un *migration act* finalmente capace di diventare atto doveroso all'interno dell'Unione europea. Mi permetto, però, di dire che molto di più si accingono a fare il sottosegretario Sandro Gozi e, prossimamente, nel Consiglio europeo, Matteo Renzi. Sta passando, infatti, sotto silenzio come l'Unione europea e l'emergenza profughi si affrontino anche attraverso atti rilevanti quali ritenere, nei fatti, le frontiere di ogni Stato che si affaccia sul mare una unica frontiera europea. Quindi, quei mari, quei

La Polizia unica di frontiera, un'unica Guardia costiera, è un avvenimento di straordinario valore, cui dare merito nella determinazione che questo Governo sta avendo. Il 6 ottobre, infatti, è stato ratificato, e nelle prossime e nelle prossime settimane verrà realizzato, questo progetto, che non è solo la certificazione di un'unica frontiera, ma anche di politiche comuni contro gli abusi, i traffici illeciti di rifiuti, i traffici illeciti di armi e di uomini, nel pieno rispetto dei dettami di civiltà che l'Europa, nel suo complesso, deve far prevalere, rispetto a interessi spiccioli o anche nazionali. Bene anche il forte potenziamento degli aiuti all'Africa, aiuti destinati a istruzione, ricostruzione e lavoro, in modo da mantenere nelle loro terre

dalle nostre frontiere verso questi mari possano far presumere anche un'Europa unita e più forte.

Presidente del Consiglio andrà a Bruxelles, a parlare principalmente di immigrazione, un tema molto complesso, che è già stato affrontato in numerosi appuntamenti senza che siano mai usciti fatti concreti. Ma volete sapere quanto conta il nostro Primo Ministro in Europa? Abbiamo fatto i calcoli. Grazie al voto del Parlamento europeo, l'Italia è riuscita a strappare un minimo di solidarietà agli altri Stati membri: il ricollocamento di 39.600 migranti, su un pacchetto complessivo di 160.000, da redistribuire proporzionalmente in tutti i 28 Paesi membri. Invece, al 30 settembre, hanno lasciato l'Italia 1.258 richiedenti asilo, appena il 3,1 per cento del totale. Altro punto della discussione saranno i trattati internazionali TTIP e CETA. Il Trattato transatlantico non è una normativa nata da un processo democratico, bensì un accordo contrattuale scritto da funzionari non eletti e non rappresentativi. Il Governo Renzi, invece, continua a sostenere con forza l'approvazione del Trattato transatlantico, dichiarandosi favorevole addirittura ad una procedura *EU only* ed esautorando gli Stati nazionali. Questo procedimento è ammissibile per i trattati economici, ma non per il TTIP, che è invece un trattato di tipo misto. In realtà, proprio l'Italia ha posizioni incompatibili con le clausole negoziate dagli americani, dovendo difendere 42 eccellenze del *made in Italy* dall'assalto dei prodotti americani. Se il TTIP oggi è in stato comatoso e passerà a miglior vita, lo si deve solo alla volontà di milioni di cittadini europei, che hanno manifestato lungamente e fortemente, costringendo i governanti europei a prenderne atto. Anche il terzo punto all'ordine del giorno, ovvero le relazioni con la Russia, il cui embargo - come abbiamo sentito - ci è costato 1,5 miliardi di euro di mancato *export*, non fa che sottolineare come il Presidente del Consiglio sia considerato in ambito europeo. Gli altri decidono, badando principalmente ai loro interessi, e noi subiamo; tanto l'unica cosa che il Presidente del Consiglio è in grado di organizzare è una minicrociera a Ventotene. Credo che il comportamento che l'Europa ha nei suoi, e conseguentemente anche nei nostri, confronti sia dovuto al fatto che il Presidente del Consiglio non è più credibile e racconta palle in quantità industriali; e per un professionista non c'è cosa peggiore che non essere credibili. Che lui sia un professionista della politica non ci sono dubbi: è passato da una carica pubblica all'altra senza discontinuità temporale. Il miglior Berlusconi l'avrebbe chiamato "fanigottone". La credibilità e l'autorevolezza del Presidente del Consiglio sono minate dalla sua propensione a raccontar palle, da quelle sulle banche ai numeri del *jobs act*,

Ci sono però numeri che sono macigni: 107.000 italiani hanno lasciato l'Italia nel 2015 (non uno zero virgola), cui si devono aggiungere i 101.000 del 2014. Questi giovani sono il nostro futuro, coloro che hanno forze e idee, che invece andranno ad arricchire gli altri Stati. Vogliamo parlare poi delle *brochure* per incentivare gli investitori esteri a venire in Italia, in cui si diceva che un ingegnere costa mediamente 10.000 euro all'anno in meno rispetto al resto d'Europa e che la crescita del costo del lavoro nel triennio 2012-2014 è stata la più bassa dell'eurozona? In questo ambito credo che solo Erode abbia fatto peggio di lui. Erode ha ammazzato una generazione, lui l'ha costretta a emigrare. Dottor Renzi, se lei ritiene che le mie parole siano esagerate, la invito a leggere non il *blog*, ma alcune testate giornalistiche internazionali indipendenti, quelle poche che lei e i suoi amici della J.P. Morgan non avete ancora comprato. Comunque, da qualunque parte lo si guardi, lo schiaffo che le ha dato qualche giorno fa Moscovici, commissario europeo agli affari economici, è portentoso e sonoro e dovrebbe indurla a una serena riflessione.

Sì, avete capito bene: se il Movimento 5 Stelle non fosse una forza politica coerente e credibile, non acquistabile, che fa paura all'Europa perché sta dalla parte del cittadino, non avrebbero concesso quella flessibilità che chiede Renzi, necessaria per comprare i voti referendari. Dottor Renzi, si ricordi che la flessibilità che verrà concessa non è dovuta alla sua bravura, ma al fatto che c'è il Movimento 5 Stelle. penso che l'Italia abbia bisogno di più Europa, anche se l'Europa è gestita in modo insufficiente da burocrati mediocri.

Ci vuole una vera politica per l'immigrazione da parte dell'Europa, tenendo conto che l'instabilità politica, le guerre, il terrorismo hanno cambiato i presupposti sui quali si basavano gli accordi precedenti. Sul piano economico dobbiamo essere credibili. Il fatto che la variazione del DEF non sia approvata dall'Ufficio parlamentare di bilancio non aumenta la nostra credibilità, anzi riduce a zero il prestigio internazionale dell'Italia. Vorrei, infine, ricordare un dato di fatto. Probabilmente otterremo flessibilità, ma dobbiamo ricordarci che la parola «flessibilità» è sinonimo di «debito pubblico», di indebitamento ulteriore. Questo significa che il debito pubblico aumenterà e ciò comporterà per le generazioni future più tasse, più problemi, meno benessere: non credo sia un grande risultato.

come gli 80 euro e ora i soldi ai pensionati - a persone che hanno il diritto di avere più soldi. Per carità, sono soldi spesi moralmente bene, ma dobbiamo prendere atto che questo tipo di spesa, da una parte, aumenta il nostro debito e, dall'altra, non migliora la situazione economica del nostro Paese e, pertanto, produce effetti molto negativi sulla situazione economica dell'Italia attuale, ma soprattutto del futuro.

Credo che oggi siamo abituati a parlare dell'Unione europea soprattutto con riferimento ai temi economici e ai margini di flessibilità del Patto di stabilità e crescita. Vorrei però ricordare che l'Unione europea ha anche un'altra dimensione, che è importante e che non dobbiamo trascurare, contenuta nei contenuta nei primissimi articoli del trattato sull'Unione europea, che riguarda i principi sui quali essa si fonda. Con il suo permesso, vorrei leggere l'articolo 2 e la prima parte dell'articolo 3, dove si afferma che «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». «L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima». Quando oggi ho sentito fare considerazioni critiche nei confronti dell'Unione europea da parte di alcuni colleghi, ho ho avuto la conferma di un sospetto che nutro da tempo: oggi chi è nemico dell'Unione europea è nemico di questi valori e chi, invece, difende l'Unione europea difende questi valori. Più volte è stato detto che ci sono dei populismi che stanno cercando di disgregare l'Unione europea, ed è vero. Abbiamo visto anche oggi prendere la parola gruppi che sono alleati nel Parlamento europeo, o che lo sono stati,

e che sono quindi nemici dei valori nei quali noi ci riconosciamo. Oggi noi abbiamo una battaglia politica che non è soltanto tra Stato e Stato ma tra chi è portatore di un certo tipo di valori e chi invece li nega, magari affermandoli in via teorica ma poi, con comportamenti ambigui e grigi, rigettandoli nella pratica. Questi sono populismi di cui oggi non abbiamo bisogno perché sono nemici della storia dell'Unione, quella abbiamo dato un contributo fondamentale (e intendiamo continuare a farlo con un'azione che è stata assolutamente pregevole del Governo italiano, che si è fatto rispettare, ha riconquistato credibilità nell'Unione europea e oggi acquista, grazie a tale credibilità, uno spazio di manovra economica fondamentale per ridare slancio alla nostra economia). Credo sia importante ciò che è stato oggi ricordato da parte del sottosegretario Gozi

un freno, una certa prudenza, ma successivamente ci siamo avviati lungo la linea che è stata indicata dal Governo italiano. Signor Presidente, vorrei brevemente ricordare alcuni punti in materia di immigrazione che mi pare siano fondamentali. Noi dobbiamo attuare il principio di solidarietà tra gli Stati membri e quegli Stati che non rispettano tale principio e non rispettano i principi contenuti nell'articolo 1 e nell'articolo 2 del Trattato vanno sanzionati come coloro che violano altri punti del Trattato. L'Unione europea deve difendere i propri principi anche quando si tratta di valori e non soltanto di parametri economici. Noi dobbiamo continuare a portare avanti un'azione che salvi le vite umane, soprattutto quando sono in pericolo e quando si trovano in mare. È un principio di civiltà cui non possiamo derogare e non possiamo accettare i comportamenti e gli atteggiamenti grigi di coloro che da una parte dicono che, sì, dobbiamo salvare i migranti, poi però li dobbiamo rimandare indietro. Ho ascoltato parole che non condivido affatto. E anche sull'atteggiamento nei confronti della Russia,

Dobbiamo certamente superare il regolamento di Dublino e chiedere ai nostri *partner* di farlo e attuare un sistema centralizzato di gestione delle domande di asilo. Dobbiamo far rispettare gli accordi di ricollocazione che sono stati assunti dai nostri *partner* e che li impegnino a ricollocare un numero di persone assai maggiore di quelle che fino ad oggi hanno accettato di ricollocare. Dobbiamo attivare dei percorsi, dei corridoi umanitari per cercare di evitare la tratta che viene svolta all'interno del Mediterraneo e aiutare coloro che sono in pericolo di vita ad avere diritto quantomeno alla sopravvivenza. Dobbiamo lottare, quindi, contro lo sfruttamento dei migranti, aprire dei canali di immigrazione economica perché non sono soltanto i rifugiati che hanno diritto a venire nel nostro Continente. Il nostro Continente è stato costruito anche grazie alle immigrazioni economiche. Molti di noi sono figli e nipoti di migranti economici di migranti economici che sono una grande risorsa per un Continente che oggi fa fatica, perché sono le persone che hanno più motivazione a essere protagoniste della ripresa economica e noi dobbiamo valorizzarle, non dobbiamo lasciarle marcire nei centri di accoglienza, nei CIE, dobbiamo sviluppare il loro entusiasmo per la vita, per l'attività economica economica e chiedere loro di aiutarci a migliorare le condizioni del nostro Paese, perché c'è tanto da fare nel nostro Paese, ci sono tanti lavori che i nostri connazionali non sono più disposti a fare. Valorizziamo queste risorse e questo entusiasmo, diamo loro accoglienza esigendo al tempo stesso che,

dobbiamo cercare di andare ad agire sulle cause dell'immigrazione, il che vuol dire avviare percorsi di *partnership* economica e di crescita con i Paesi di origine dei migranti, avviando con più decisione un'azione sul piano della cooperazione internazionale che aiuti questi Paesi a creare le condizioni per le quali, poi, la migrazione possa essere regolamentata con dei flussi più accettabili e più pianificati di quanto siano oggi, perché oggi il problema non sono i flussi ma la situazione assolutamente caotica nella quale si muovono questi migranti.

Questi sono i valori nei quali, come Partito Democratico, ci riconosciamo e per i quali siamo disposti a fare delle battaglie forti, a testa alta, senza vergognarci assolutamente di ciò che abbiamo fatto in questi anni. *(Applausi

e impegni che l'Unione europea oggi ha assunto e che - come lei sa benissimo - sono parole e impegni che prima parlavano solo italiano e sono del tutto attribuibili, a partire dal semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea, all'azione del nostro Governo. Vorrei ricordargliene alcune:

infatti, giustamente, avete più volte chiesto all'Italia - e, attraverso il nostro Governo, all'Europa - di cambiare l'approccio sul tema dello sviluppo e dell'immigrazione innanzitutto rispetto all'Africa. Giustamente avete sempre sostenuto che l'Africa deve essere la grande priorità europea. Noi ci siamo battuti per questo oggi stiamo negoziando dei patti sulla migrazione che devono combinare una nuova strategia di investimenti pubblici e privati, per i quali la Commissione europea si è impegnata a stanziare risorse. Nella valutazione del presidente Juncker queste risorse arriveranno fino a 44 miliardi di euro - per noi si deve andare anche oltre, ma è importante avere un nuovo strumento - che si aggiungono al bilancio attuale, in cambio di impegni, da parte dei Paesi di origine, ad affrontare insieme a noi le cause principali dei fenomeni migratori: un insufficiente sviluppo, ma anche la lotta contro i trafficanti di esseri umani e contro traffici di vario genere. Questo è quanto stiamo facendo

anche nostra - e avete sentito il Presidente del Consiglio ribadirlo più volte in quest'Assemblea - il presidente Juncker e la Commissione europea si sono impegnati a raddoppiare quel Piano, tenendo presenti alcune grandi priorità come l'ambiente, il digitale, le piccole e medie imprese, arrivando a mobilitare fino a 630 miliardi di euro, rispetto ai 315 iniziali, da qui al 2020. Questa è un'altra risposta concreta che va nella direzione che tanti Gruppi hanno auspicato, ed è la direzione nella quale vuole andare l'Italia. Consideriamo questo sufficiente? No.

Romano Prodi aveva ragione quando definì il Patto di stabilità stupido se applicato in maniera rigida. Oggi abbiamo un Presidente della Commissione europea che si è impegnato ad attuare una regola, quella della flessibilità, che vuol dire applicare il Patto di stabilità in maniera intelligente. Credo che quando c'è un commissario che conferma questa linea, tutte le forze politiche dovrebbero dire: «Bene, finalmente un fatto di buon senso, un passo in una buona direzione», anziché

Ritengo importante invece impegnarsi insieme - lo diceva la senatrice Puppato - per assicurare che i passi in avanti compiuti vengano finalmente tutti attuati; quindi, è certamente molto importante che sia subito operativo il Corpo di polizia europea e la Guardia costiera delle frontiere esterne, perché quella è la risposta europea che vogliamo. Non sbagliamo obiettivo in materia di frontiere: la risposta per gestire il tema dei flussi umani e anche la sicurezza non è stabilire le frontiere tra Italia e Austria o tra Italia e Francia, non è tornare alle frontiere nazionali, ma è lavorare insieme con strumenti comuni e con impegni veramente europei, là dove c'è la necessità di intervenire, cioè le frontiere esterne. Da questo punto di vista crediamo che questo sia un passo in avanti molto importante. Sono d'accordo con quanto diceva il senatore Barani sull'insufficiente rispetto degli accordi di distribuzione dei richiedenti asilo.

queste sono alcune considerazioni che ritenevo importante fare. Adesso, se lo consente, passo ad esprimere i pareri sulle

il parere è contrario ai primi tre e favorevole agli ultimi due. Per quanto riguarda la risoluzione n.

Signor Presidente, ovviamente il nostro Gruppo è grato all'onorevole Gozi per come ha riassunto stamattina il discorso del Presidente del Consiglio alla Camera

è Bratislava. E no! Prima di Bratislava, il Governo aveva dato appuntamento alla comunità internazionale, alla memoria storica dell'europeismo italiano, a Ventotene. Quindi, le premesse erano ben diverse da quella conferenza stampa di Bratislava che ha portato poi - lo capisco - l'onorevole Gozi

un partito d'opposizione che ha il senso dello Stato nazionale e della politica internazionale condivisa e, quindi, accettiamo l'invito del Presidente del Consiglio a condividere sempre di più; però, affinché si possa condividere, è necessario un tasso di personalizzazione della politica estera un po' meno spinto e un po' meno spregiudicato di quello

Ieri sera, nella discussione sul calendario, un collega che ha molto prestigio su tali questioni, il senatore Mario Mauro, ha ricordato come in molti Paesi d'Europa, soprattutto in Germania,

Questo è fisiologico della politica nell'accezione moderna, ma da questo punto di vista, mi si consenta di rilevare che, da parte del Presidente del Consiglio, ne è fatto sempre più uso e abuso. Veniamo a qualche punto più specifico. Sulla questione dell'emigrazione sfugge al Governo italiano come proprio il Governo tedesco e la cancelliera Merkel organizzato un proprio viaggio nel Mali, nel Niger e nell'Etiopia, e cioè in quei Paesi nei quali il Presidente del Consiglio ha annunciato questa mattina il negoziato per aprire canali diplomatici. A parte il fatto che questa minaccia formulata nelle conferenze stampa di Bratislava del presidente Renzi - ma anche, più di cent'anni fa, nei momenti importanti dell'unità nazionale - che l'Italia farà da sé non ha mai portato grande fortuna al nostro Paese, stiamo attenti e assumiamo anche un atteggiamento critico, ma attenzione al nazionalismo. Visto che sto affrontando il tema, ne parlo a proposito di un grande Paese democratico, la Gran Bretagna. un'accidiosa intransigenza nazionalista. Abbiamo sentito circolare proposte come la limitazione degli studenti stranieri o, addirittura, l'esigenza di far sapere il numero dei dipendenti non inglesi da parte delle aziende. Beh, da questo punto di vista, ci attendiamo

Tanto più che proprio il Presidente del Consiglio ha citato stamattina un grande europeista di tradizione socialista, Jürgen Habermas, il quale ha parlato di frenetico immobilismo dell'Europa. Il frenetico immobilismo dell'Europa certamente esiste, ma se posso anch'io personalizzare a fini di spersonalizzazione, anche il renzismo - questo modo di partecipare alla conferenza stampa con un vestito e al Consiglio con tutt'altro vestito dell'attuale Presidente del Consiglio - è frenetico immobilismo. È un frenetico immobilismo che dobbiamo correggere. Anche per questo, senza senza pregiudizio di altri atteggiamenti, noi ci asterremo sulla risoluzione di maggioranza. Ci asterremo anche sulle altre risoluzioni. Possiamo forse votare a favore della nostra, anche se, come ho spiegato, condividiamo, ma non possiamo

Il vertice prevede anche, sia pure come inizio di discussione, un dibattito sul rapporto con la Russia. Il vertice è domani. Sono quattro o cinque giorni che in Germania e in Francia non si parla che di questo. A me sembra che l'avarizia di considerazioni in materia del Presidente del Consiglio nel Parlamento italiano faccia parte di quel tatticismo tanto ben documentato ieri sera dall'onorevole Mauro Mario. A maggior ragione, grati all'onorevole Gozi, formuliamo un nostro voto complessivamente di astensione.

abbiamo assistito in Aula a un dibattito tranquillo, moderato e dai toni pacati, contrariamente a quanto è successo alla Camera dei deputati, dove il Governo ha mandato un'altra persona che - ahimè - ha deciso di togliere i panni del Presidente del Consiglio e trasformarsi in in istigatore, lanciando strali e insulti a tutti coloro che si oppongono alla sua marcia trionfale verso il 4 dicembre. 4 dicembre. Ieri avevamo detto che lo avremmo voluto in Aula; ben venga invece avere lei, onorevole, piuttosto che il Presidente del Consiglio, cui io mi rivolgerò. Per me era infatti necessario averlo in Aula per potergli riferire quello che noi pensiamo. la flessibilità, onorevole Presidente, sappiamo tutti come sta funzionando. Visto e considerato in Europa ci sono i populisti brutti un po' di soldi. Pertanto, 19 miliardi di euro di flessibilità nei due anni precedenti e adesso ne arrivano altri 7: debiti su debiti. L'Italia continua quindi ad indebitarsi per far fare al presidente del Consiglio Renzi bella figura in vista del *referendum* del 4 dicembre. Sull'immigrazione, colleghi e Presidente del Consiglio assente, non intervengo. Lo dico molto onestamente. Non interveniamo perché tutte le volte abbiamo sempre detto e fatto

Ricordiamo solamente dei numeri e lo facciamo per lasciarli alla memoria dei posteri, dei prossimi senatori eletti che arriveranno in quest'Aula; 144.518 sbarchi. Per quanto riguarda l'accoglienza siamo messi peggio, perché nel 2013 eravamo a 22.000 persone accolte - e quindi aiutate

Quando diciamo che l'immigrazione, in questo caso molto spesso clandestina, è un *business* per qualcuno, lo diciamo a ragion veduta. Tra qualche

Per quanto riguarda tutto il resto, caro presidente del Consiglio Renzi, partiamo dal tema a lei più caro. Non mi riferisco infatti ai problemi dell'Italia, ma al *referendum* costituzionale. Nella storia della Repubblica non si era mai visto un Presidente del Consiglio a cui fosse venuta l'idea di personalizzare un *referendum* costituzionale. Non crediamo che sia così ingenuo da aver fatto un errore, come va in giro a dire adesso.

A nulla vale il fatto che il consulente di immagine, pagato da tutti noi, il signor Messina, nel formare i volontari che gireranno per indottrinare alle ragioni del sì, continui a dire di non legare il *referendum* al Presidente del Consiglio.

Quindi, ricordiamo al Presidente assente - sempre assente - che durante il suo Governo la più grande azienda italiana, la FCA, ha preso armi e bagagli ed è andata all'estero, trasferendo la sede: non male! Lei mi dirà, signor Presidente del Consiglio,

Non può mancare anche una riflessione sull'Europa, visto che domani ci andrà: adesso è molto più chiaro perché continua a farci restare servi della Merkel. Lei sostiene che, se l'Italia uscisse dall'Europa, lo *spread* schizzerebbe in alto. Presidente assente, ci spieghi come mai, durante i suoi due anni e mezzo di Governo, sebbene lo *spread* sia a livelli bassissimi, il debito pubblico è in continuo aumento? Ciò avviene perché siete degli spendaccioni,

tutte scuse quelle che lei va dicendo, affermando che non si può governare con due Camere: lei non è in grado di governare. Infatti, con mille giorni ha avuto tutto il tempo e poteva dimostrare qualsiasi cosa, invece non è stato in grado di fare niente: non è stato in grado di risollevare l'economia di questo Paese, non è stato in grado di rispettare le promesse fatte agli italiani. Le chiediamo una cortesia: eviti eviti di spacciarsi per esperto finanziario. Magari si potrà spacciare per esperto in inglese, ma non per esperto finanziario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. A luglio lei diceva che bisognava investire comprando le azioni della banca Monte dei Paschi di Siena,

Non è bastata Banca Etruria? Ora c'è Monte dei Paschi. Per caso, pur di far vincere il sì al *referendum* è disposto a tutto? Abbiamo sentito che due banche americane, Goldman Sachs e JP Morgan, si sono schierate per il sì. Scusi, Presidente, JP Morgan è la banca che sta sistemando il *dossier* della banca Monte dei Paschi di Siena? Dare per ricevere: lei propaganda di comprare azioni della banca Monte dei Paschi e loro dicono che al *referendum* è giusto votare sì. Il Partito Democratico non faceva parte di quelli che dovevano aiutare i più deboli? Oggi, invece, sta aiutando le banche, che sono tutto tranne che soggetti deboli.

degli italiani che credevano in lui e che purtroppo in questo momento sono rimasti fregati. Le porto due esempi: il signor Alessandro e il signor Fabio. Il signor

che si è suicidato: era un vigile del fuoco precario che è stato licenziato e si è tolto la vita. Questo, signora Presidente, è un omicidio di Stato, perché sono anni che i vigili del fuoco precari chiedono a a questo Governo, a quello precedente e a quello ancora prima di essere sistemati, ma non stanno ricevendo risposte. Sono qua a portare la voce del signor Fabio e di tutti i suoi colleghi che qualche giorno fa erano davanti a Montecitorio a protestare. In quell'occasione tanti colleghi del Partito Democratico sono andati a riempirsi la bocca a riempirsi la bocca e a fare promesse: risolvete i problemi degli italiani e poi parleremo della Costituzione.

una risoluzione Zanda, Schifani, Zeller, del 16 marzo 2016; oggi, un'altra risoluzione con i due terzi dei nominativi assolutamente identici e, probabilmente, con l'efficacia che

Lo ricordava il senatore Centinaio: siamo a mille giorni di Governo ma, soprattutto, siamo ormai a decine di dibattiti e impegni assunti da questo Governo rispetto alle problematiche enunciate dal sottosegretario Gozi.

Non può esistere un Governo che insegue gli impegni futuri senza mai dover dar conto, anche da un punto di vista morale, degli stati degli stati di avanzamento rispetto al programma di lavoro che si era dato. Cosa volete dire a quei parlamentari di maggioranza che hanno votato favorevolmente alle precedenti mozioni a firma Zanda, Schifani, Zeller, oggi Zanda, Bianconi, Zeller? Cosa volete dire rispetto al parere favorevole che avete espresso? A quel voto di maggioranza? Metto da parte anche il ruolo, che potremmo giocare oggi, delle facili Cassandre, quando vi dicevamo che le vie di uscita rispetto a quei problemi erano altre, altre, esortandovi a assumere impegni diversi, ma rispetto ai vostri impegni, ai vostri voti, alla vostra azione di Governo. Ma cosa venite a dire oggi? Quale altro voto chiedete alla vostra maggioranza, senza neanche sviscerare gli aspetti critici? La verità è una sola, e avreste dovuto avere il coraggio di declamarla oggi nei due rami del Parlamento. Abbiamo bisogno di recuperare prestigio e credibilità in Europa. Da questo punto di vista il Governo Renzi ci ha fatto fare enormi passi indietro.

Sottosegretario, nel suo intervento iniziale, a discutere e a dare indicazioni rispetto al bilancio pluriennale dell'Unione europea. Ma è un bilancio dove voi non esercitate neanche il minimo della *moral suasion* e della pressione. Altro che utilizzare il diritto di veto per l'Italia! Voi prendete atto di decisioni che vengono assunte presso la Cancelleria tedesca; prendete atto di decisioni assunte presso la Cancelleria tedesca e appena condivise con la Francia per poi venire a contrattare, rispetto al bilancio della Comunità europea, soltanto quello che vi interessa dal punto di vista propagandistico a livello interno: la possibilità di indebitare ulteriormente lo Stato italiano per poter fare le campagne elettorali che purtroppo sono in corso. Ma vedete quanto ci sta costando questo *referendum* del 4 dicembre? Vedete quanto tempo perso, quanto lavoro da fare per l'Italia che invece viene dirottato, con tutte le energie del Governo? Vi Vi vediamo tutti in giro, Ministri, Sottosegretari, più o meno dirigenti di partito, tutti buttati in giro solo per una cosa, la madre di tutte le battaglie: il *referendum* costituzionale. Ve ne fregate del bilancio pluriennale della Comunità europea. Ve ne fregate dell'esercizio del bilancio e della legge legge di stabilità nazionale e soprattutto ve ne fregate di un fatto, caro sottosegretario Gozi: lei oggi ha la responsabilità morale di ulteriori 140.000 sbarchi sulle coste europee. Lei oggi si assume la responsabilità morale, a nome del Governo, del fallimento totale e assoluto delle politiche sull'immigrazione. tratta di un fallimento totale e non avete un solo punto da portare a vostro vantaggio, se è vero che ne sono morti altri 3.500 nel Mar Mediterraneo. Collega Cociancich, non è un problema di diversa sensibilità.

assumono accezioni negative solo quando sono esasperazioni di sentimenti che non sono condivisi a livello sociale. Quando invece ci si fa bandiera rispetto a un malessere, a un disagio,

rispetto a dei problemi che non possono essere affrontati con delle risoluzioni che rimangono sulla carta e che non hanno nessun riscontro. E cosa dirvi degli impegni dei precedenti Consigli europei rispetto alle popolazioni produttive? Ancora aspettiamo Gozi che ci venga a dire della messa in mora rispetto a dei trattati europei per quanto riguarda gli scambi commerciali nel Mediterraneo. Che cosa avete ancora da dire rispetto alle tante risoluzioni approvate? Richiamo all'attenzione i colleghi della maggioranza: essere di maggioranza non significa soltanto essere obbedienti, ma significa anche avere la forza di far passare le proprie idee. Voi stessi, che vi siete espressi più volte contro la concorrenza sleale dei trattati economici, oggi ci dite che il Trattato con il Canada, che tra l'altro è sotto giudizio della Corte di giustizia europea, diventa una nuova frontiera. Ma fate piuttosto delle verifiche rispetto alle nostre associazioni produttive e rispetto ai nostri mondi.

del Regno Unito dall'Unione europea. Ma si preoccupi invece dei giovani italiani. Si preoccupi di quei tanti giovani che stanno abbandonando il nostro Paese per raggiungere l'America o l'Australia. Si preoccupi di quelli che non hanno neanche avuto la possibilità di dire mi piace o non mi piace, ma sono stati costretti dalle esigenze di lavoro a lasciare il nostro Paese! Per questi giovani cosa avete fatto? Cosa avete sbattuto sul tavolo dell'Europa? Il grande piano Juncker. Ha relazionato il Governo in Assemblea sullo stato di attuazione del piano Juncker?

siete oggetto di attacco o di critiche profonde. Siete oggetto della nostra riprovazione e della nostra contrarietà perché siete assolutamente inefficaci signora Presidente, per il termine che sto per utilizzare - inutili rispetto alla soluzione dell'Italia. Siete assolutamente inadeguati voi, non per un fatto ideologico, di contrapposizione, ma perché, rispetto a quello che promettete nelle varie proposte non riuscite a portare alcun risultato. Signora Presidente, vedo che per fortuna abbiamo risolto il problema della proposta di risoluzione che non risultava agli atti e il Sottosegretario ha così immediatamente potuto esprimere il parere.

Per quanto riguarda il discorso in generale, penso che il Consiglio europeo cui ci apprestiamo assuma un carattere molto probabilmente interlocutorio, anche per il anche per il tipo di argomenti che affronta. Tra questi ce ne sono alcuni che hanno un carattere immediato, come quello sull'immigrazione, ma ce ne sono altri maggiormente

Purtroppo oggi dobbiamo constatare un atteggiamento da parte dell'Unione europea che rallenta le questioni che devono essere affrontate. sul problema dell'immigrazione dobbiamo constatare un ritardo pesante da parte dell'Unione europea e bene ha fatto l'Italia a smuovere le acque. Non per niente, proprio oggi e in questi giorni, attraverso - ad esempio - la visita in alcuni Paesi dell'Africa da parte di *leader* di altri Paesi europei, si sta ribadendo l'utilità

come non può rimanere insensibile l'Europa attraverso una politica di disattenzione e di mancanza di rispetto nei confronti dei presupposti del nostro stare insieme, tra cui quello di assumerci, tutti insieme, le responsabilità di fronte a questo problema epocale. Allora ben venga la nuova Guardia costiera europea che va a sostituire l'esperienza di Frontex. Speriamo che questa

Ecco allora la necessità di una rivisitazione del Regolamento di Dublino, come è stato ricordato dal Sottosegretario.

noi speriamo che dal prossimo incontro del Consiglio europeo, che avverrà in questi giorni, venga uno slancio nuovo, uno slancio diverso, e che si sappiano affrontare anche temi importanti come quello della

Sono aspetti importanti che vanno sottolineati, tenuti presenti e valutati nella loro realtà. Per quanto riguarda l'aspetto commerciale, il Sottosegretario ci ha chiesto di espungere dal nostro ordine del giorno una frase. Lo facciamo volentieri, ma ciò non

con un riferimento - com'è stato fatto anche da altri colleghi e come abbiamo fortemente sottolineato nell'ordine del giorno - ai rapporti di una politica intelligente nei confronti della Russia.

colleghi e colleghe, onorevoli rappresentanti del Governo, ringrazio innanzitutto il sottosegretario Gozi che nella sua replica ha manifestato la volontà del Governo di affrontare, in vista dell'imminente viaggio negli USA del presidente Renzi, la vicenda di Chico Forti. Come ho già detto in discussione, senza l'Europa il mondo è meno stabile e sicuro. Senza l'Europa ciascun Paese diventa più debole e fragile, non in grado di misurarsi con la complessità di questo nostro mondo. L'Europa deve arrestare la corsa alla demolizione, frutto degli egoismi nazionali, per tornare a essere il luogo della speranza, il punto dì riferimento per le generazioni del futuro. Ciò che il Governo ha posto, anche in riferimento agli obiettivi del Documento di bilancio,

quale unico ambito strutturale e globale che possa rendere compatibili e sostenibili gli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto del quadro di compatibilità, in riferimento al quale il nostro Paese non ha richiesto alcuna deroga. Non comprendere, in Italia e in Europa, come in una fase di recessione finanziaria ed economica di assoluta gravità non vi siano opzioni alternative a una revisione dei meccanismi e degli obiettivi di governo della finanza pubblica, al fine di evitare una visione delle politiche di bilancio che potrebbe avere conseguenze distorsive anziché favorire il rispetto degli obiettivi di saldo strutturale, equivale a porre in discussione la stessa sopravvivenza delle istituzioni europee e a incrementare le politiche di chiusura che determinano, già oggi, e ancor più possono produrre, una significativa riduzione della capacità europea di essere soggetto unitario e competitivo in grado di affermare - come è riportato nella risoluzione di maggioranza che abbiamo sottoscritto e che sosteniamo - una nuova *governance* europea. Dice bene il sottosegretario Gozi quando afferma che il Patto di stabilità o viene applicato con intelligenza o semplicemente è stupido. Anche per questo, auspico un intervento del Governo per risolvere la vicenda dell'avanzo di bilancio della Provincia autonoma di Trento, cui ho accennato in discussione generale. annuncio che il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE voterà a favore della risoluzione n. 3 di maggioranza, a prima firma Zanda e sottoscritta anche dal presidente Zeller a nome del nostro Gruppo. È una risoluzione molto precisa e articolata che affronta tutti i nodi sul tappeto, ma soprattutto la crisi economica e ideale dell'Unione europea, per rilanciare l'intuizione iniziale e affrontare seriamente e con determinazione il problema dell'immigrazione, i cinque *compact* con i Paesi africani prioritari, il controllo dei flussi, i rapporti con la Russia, con la Cina e gli Stati Uniti, la revisione del TTIP, la crisi ucraina e la Brexit.

sempre ai fini della campagna referendaria a favore del «sì». Qui, invece, il sottosegretario Gozi ha tentato di fare una relazione che entrasse nel merito delle questioni che sono di fronte a noi al Consiglio europeo. Questa situazione francamente è imbarazzante. Lo dico con molta tranquillità: vi pare questo un modo di prepararsi al Consiglio da Paese serio? Penso che ciò non accada in nessun altro dei Paesi dell'Unione europea e francamente fa parte della stessa modalità che ha accompagnato tutta la vicenda di Bratislava. Ciò è tanto vero che gli altri *partner* europei ci hanno tenuto a far sapere che l'Italia aveva firmato, ma fuori il presidente Renzi ha pensato bene, a uso e consumo di chi ci vuol credere, di fare le sceneggiate contro.

utilizzate per investire nelle politiche di sviluppo e di crescita, in un piano investimenti, e questo fa il paio con le critiche che il mio collega giustamente ha fatto anche alle prese di posizione del commissario Moscovici, il quale addirittura dice: «Sì, io vi sostengo, vi do flessibilità», ma non per dire che si faccia un piano di investimenti, si investa con risorse in modo strutturale per accompagnare la crescita; noi oggi presenteremo il nostro *social compact*, ad esempio, con una serie di proposte». No, dice: «Io vi posso al limite aprire sulla flessibilità perché vi devo sostenere nella campagna referendaria». Questo non l'ha detto esplicitamente. Forse si potrebbe

Sottosegretario, lei ha visto

completamente e totalmente la questione posta, su cui tutti unanimemente avevamo detto che bisognava chiedere e pretendere una modifica. Lo stesso si può dire per quanto riguarda il piano di riallocazione.

sia per quanto riguarda il Canada che per quanto riguarda il TTIP. Per questo motivo non possiamo accettare le sue proposte di riformulazione.

Sottosegretario, fa un lavoro ai più sconosciuto, segreto e sotterraneo, ma preziosissimo. Lo sappiamo e gliene vogliamo rendere merito. Lei ha una conoscenza e una stima in Europa

alcune brevi parole per dire che noi approviamo la relazione fatta dal sottosegretario Gozi e abbiamo sottoscritto convintamente

Credo che l'Europa dovrebbe farsi carico di quello che desiderano i cittadini, che forse sono più lungimiranti dei loro governanti.

ha citato una frase, che condivido, ma non si riferisce al suo discorso: ha detto che l'Europa è una *summa* di riassunti. Ogni riunione europea non è altro che un riassunto dei riassunti precedenti.

La crisi siriana è una delle più complicate degli ultimi decenni. Non ho mai sentito un rappresentante del Governo italiano parlare con compiutezza e conoscenza della crisi siriana. Non ho mai sentito parlare dell'osservatorio siriano dei diritti umani e non ho mai sentito parlare nei termini in cui è questo osservatorio: è un signore che abita a Coventry da circa diciotto e lavora nel negozio di abbigliamento di sua moglie e che nulla sa di ciò che accade in Siria. Purtuttavia, è la fonte di informazione più precisa e puntuale di tutte le agenzie e i *media* occidentali sulla crisi siriana. Non ho mai sentito il ministro Gentiloni o il presidente del Consiglio Renzi parlare del fenomeno dei *white helmet*, che alcuni vorrebbero portare ad avere il premio Nobel. Se andate però su Internet a vedere le foto di questi protagonisti, noterete che molti di loro hanno armi in mano e si prodigano nella cosiddetta ribellione al Governo Nessuno si è mai posto il problema di chi siano esattamente i ribelli siriani. Sono quelli di al-Nusra, camuffati con un'altra sigla, o sono veramente ribelli che hanno come vocazione naturale l'instaurazione di un regime democratico? E quindi, quando si parla di *summa* dei riassunti o di genericità della risposta dell'Unione europea, mi riferisco tranquillamente anche alla posizione del Governo italiano. Ma è sulla politica europea nel suo complesso che noto una manchevolezza e una carenza spaventose. Abbiamo assistito alla sceneggiata di Ventotene: Renzi è riuscito a portare sulla nave Garibaldi Hollande e Merkel - quest'ultima notoriamente soffre il mare e, quindi, non è venuta volentieri - e dopo abbiamo assistito a un incontro personale del presidente del Consiglio Renzi nella sede della Ferrari. Dopo di che ci siamo resi conto di quanto l'Italia sia esclusa dai posti di comando dell'Europa, perché nel frattempo la cancelliera Merkel ha chiesto agli Stati del cosiddetto Gruppo di Visegrád di fare un incontro in Austria e non in Lituania sulle

Ma la Germania ha anche altri problemi: non ha solo quello di rappresentare il Paese egemonico e dominante in Europa; ha un *surplus* commerciale del quale non si parla mai; ha delle banche come la Deutsche Bank, che ha circa 52.000 miliardi di derivati, che sono una bomba ad orologeria nel sistema economico europeo.

con il quale la Germania in quell'occasione, sulla nave Garibaldi e nelle nostre acque territoriali, aveva intenzione di parlare con il Governo italiano del futuro dell'Europa. Come cambiare l'Europa, come arrivare a quel famoso sessantennale dei Trattati di Roma del marzo dell'anno prossimo? Parlando e cominciando a parlare. Ho l'impressione - mi hanno detto - che di questo non si è parlato, che l'Italia in quella sede abbia fatto una figura muta e che il Presidente del Consiglio non abbia garantito al nostro Paese quel ruolo che in quella sede avrebbe potuto garantire. Mi piacerebbe sapere la verità, perché tutto ciò che è accaduto dopo sembra denotare la carenza di discussione, di approfondimento e di confronto che in quella sede sarebbe potuto avvenire. Sono pronto però ad essere smentito; lo dico nell'interesse del mio Paese.

Il presidente del Consiglio Renzi ha ricordato stamattina che la Germania ha già accettato 1.100.000 rifugiati, in questo caso, perché non sono immigrati economici. Purtuttavia, abbiamo un problema: dobbiamo bloccare l'immigrazione; e su questo punto non c'è mai una parola. C'è sempre il problema del dopo, non c'è mai il problema del prima. Noi alle volte, certi giorni, andiamo a prenderci un Comune italiano di 6.000 abitanti che viene dall'Africa per ricollocarlo in un posto che immagino sia sul nostro territorio e non andiamo mai ad impedire che questo possa avvenire. Andiamo a prelevare gommoni che sono chiusi in un *hangar*, in un magazzino che sappiamo esattamente dove si trova, sulle coste libiche, senza intervenire e avendo la capacità e la forza di farlo, perché siamo comunque presenti in Libia in misura sufficiente per fare questo tipo di intervento. Eppure, non passiamo nemmeno alla fase 2 di EUNAVFOR Med. Non abbiamo neanche la voglia, il coraggio, la decisione politica di entrare nelle acque libiche; e allora - non dico che il modello australiano sia quello da attivare - non si mettono nella possibilità di bloccare non più i barconi, perché ora sono gommoni, che hanno un'autonomia di 10-12 miglia. Arrivano le navi europee, li prendono, li imbarcano e ce li portano sulle coste italiane. C'è poi un altro problema: la circolare

declinare le impronte digitali. È però un'esortazione, non è un obbligo; e il poliziotto, secondo voi, oggi si mette nelle condizioni di obbligare qualcuno che non vuole

Mi ha colpito un passaggio questa mattina dell'intervento del Presidente del Consiglio in cui ha parlato degli Stati Uniti. che noi siamo dalla parte degli Stati Uniti nella visione del mondo perché pensiamo ai valori di libertà e di lotta contro la paura e contro una visione catastrofica del futuro incapace di dare alla democrazia un ruolo anche per il domani; che questo tipo di sguardo sul mondo sia uno sguardo che noi condividiamo profondamente. Cosa vuol dire, sottosegretario Gozi? Stiamo dalla parte degli Stati Uniti anche quando sbagliano? Siamo sicuri che dobbiamo sempre stare dalla parte degli Stati Uniti anche quando fanno errori macroscopici?

Avete sentito le cose che si sono detti i due candidati? Avete avuto percezione della inadeguatezza culturale e conoscitiva che hanno anche i candidati alla Presidenza degli Stati Uniti rispetto a problemi che noi dovremmo conoscere meglio? Quindi, prima di dire che siamo

per contraddire uno sconosciuto oratore filippino, tale Lorenzo Sumulong, prese una scarpa, o sua o del Ministro sovietico degli esteri di allora, Gromyko, e la sbatté sul banco delle Nazioni Unite. Bene, penso che Kruscev dei meriti storici li abbia anche avuti perché nel febbraio del 1956, al XX Congresso del PCUS, smontò per nostra fortuna lo stalinismo e inaugurò una nuova stagione del comunismo sovietico. Non portò certamente la democrazia: ci pensò qualche anno più tardi, parzialmente, Gorbaciov, e non ci pensava certamente Kruscev, che ebbe però un merito storico straordinario. Penso che il Presidente del Consiglio una scarpa in Europa possa anche batterla,

imprenditori del settore dei calzaturifici ma, se vuole, gliela possiamo prestare anche noi. Quindi, caro Presidente, batta una scarpa in Europa, per contraddire e contrastare gli scarponi tedeschi.

coerenza, è la politica estera. Sulla politica estera abbiamo tenuto una linea di coerenza. Lo dico al senatore Romani, che ha fatto un intervento molto dotto

Qualche volta si sa che si sta dalla parte che è più consona ai nostri interessi, ai nostri valori, al nostro modo di vedere le cose, alla nostra idea di democrazia e anche di confronto politico.

ma temo che sia una crisi profonda di quei valori che il senatore Cociancich ha ricordato come valori fondativi dell'Europa, che sono valori di solidarietà, di democrazia, di Stato sociale e di integrazione, ovvero quei valori positivi che hanno fatto

C'è un invecchiamento delle coscienze più che delle popolazioni, c'è un invecchiamento della cultura europea più di quanto dimostri l'invecchiamento demografico. C'è l'invecchiamento di una cultura che è rimasta arroccata a un periodo in cui si cercava di stare con una potenza o con l'altra, e anche questo dibattito lo dimostra. Siccome mancano le potenze contrapposte,

Dal punto di vista generale, quella che stiamo affrontando con questo Consiglio europeo è una situazione di difficoltà dell'Europa

rispetto al fatto che c'è una forte destabilizzazione e che le politiche di stabilizzazione faticano ad affermarsi e, contemporaneamente, c'è una forte divaricazione tra condizioni economiche molto forti in un mondo che cresce economicamente e condizioni economiche molto deboli in un mondo che diventa economicamente Le migrazioni sono importanti per noi ed è importante che l'Europa dia impulso ai rapporti con l'Africa e allo sviluppo di un suo partenariato di ampio respiro con Paesi africani basato sui *compact,* che consenta la gestione strutturale dei flussi migratori e non si limiti solo ad accrescere i rimpatri, pena la perdita di ogni credibilità di queste politiche. Nella proposta che andiamo a discutere nel Consiglio europeo si parla di Guardia costiera e di frontiera europea. È un passo avanti della nostra politica di tutela dalla migrazione pericolosa, della nostra politica di gestione dei flussi migratori.

è un atto concreto. Mi dispiace tanto perché le storie che si vanno raccontando mettono in secondo piano la grande nobiltà del nostro Paese e dei Paesi mediterranei come la Grecia. Mi riferisco al fatto che abbiamo messo al primo posto del nostro intervento,

ribadire la necessità di un'azione europea sui rimpatri e prevedere un richiamo alla riforma del sistema di Dublino, così come andremo a fare al vertice europeo, sono punti che mettono in campo una responsabilità, nostra ma anche collettiva dell'Europa. Si può parlare d'altro, quando non si conosce l'argomento di cui si parla, ma su questi argomenti non si può scherzare facendo della propaganda interna e ad uso interno.

degli investimenti e dell'industria ed è esattamente quanto Juncker ha sostenuto insieme al Governo italiano. I temi su cui sarebbe importante che il Consiglio europeo ribadisse la necessità di progressi concreti sono quelli degli investimenti interni (il cosiddetto piano Juncker 2.0), della lotta alla disoccupazione giovanile e del completamento del mercato unico. mercato, infatti, tende a non essere più unico e tendono a nascere frontiere per i migranti che diventano frontiere per le merci e gli scambi. E tutto questo mette in moto un meccanismo che ci riporta indietro di cent'anni, come forse la cultura politica di tanti qui. Ci riporta indietro di cent'anni e ci fa riconoscere i venti di guerra del 1914: è un meccanismo di frontiere e di steccati, ma è un meccanismo pericoloso per la pace oltre che per l'economia.

si dica che la Cina deve rispettare, nello scambio, le regole del WTO, le regole del mercato degli scambi. Dobbiamo sapere che il WTO è in una fase di crisi notevole e che questa crisi è un

e concludere la trattativa con il Canada, così come andare avanti con gli accordi sul libero scambio con il Giappone, e poi con il TTIP e con la politica atlantica, è un dovere che abbiamo verso le nostre imprese, prima di tutto, verso il nostro Paese e verso la nostra economia. Altrimenti, parliamo di imprese che non si conoscono, di mercati che non sappiamo cosa siano di mercati che non sappiamo cosa siano e di questioni che, francamente, bisognerebbe affrontare in altro modo. Vengo all'ultima questione, che ha a cuore questo vertice, ed è la questione della Russia in relazione alla crisi siriana, in relazione al fatto che si è rotto l'accordo con gli Stati Uniti d'America e che l'Italia è sempre stata per una posizione negoziale ragionevole e di mediazione attraverso le Nazioni Unite. Voglio ricordare, tra le varie cose intelligenti dette dal senatore Romani, che si è verificato un piccolo incidente sulla strada per Aleppo: un convoglio delle Nazioni Unite con 24 camion di aiuti è stato bombardato dalle batterie di Assad,

riguarda la pace di tutto il mondo e di tutto lo scacchiere, nel quale si giocano interessi molto complicati, molto più complicati di quelli che si vorrebbero risolvere mettendo in campo schieramenti contrapposti. Dovremmo portare l'Europa ad avere

aveva ricominciato a giocare un ruolo di grande potenza. Chi guarda al multilateralismo deve sapere che la Russia è una pedina fondamentale del multilateralismo,

deve farlo soprattutto l'Unione europea, aiutando gli Stati Uniti d'America in questa azione. I temi che sono in discussione al Consiglio europeo, caro Sottosegretario, sono importanti.

(senza usare le scarpe, ma usando l'intelligenza, come è più opportuno fare) di far sì che l'Europa torni ad essere quella che i suoi valori fondamentali avevano deciso dovesse essere. *(Applausi